esaminare in sede referente il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

di Consob, Banca d'Italia e Ivass, che ringrazio per la disponibilità e i contenuti proposti. La Commissione finanze e tesoro è stata chiamata ad esaminare in sede referente il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. Il disegno di legge intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858, Capo I, dalla prima alla sesta sezione, ed introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech, Capo I, Sezione VII. sezione del provvedimento contiene le disposizioni finanziarie e finali. Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito, di cui le criptoattività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle criptoattività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE va incontro al cosiddetto fenomeno di tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o alle emissioni di categoria di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito. In estrema sintesi, un registro distribuito è un *database*, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre *blockchain* nelle quali il processo di validazione non è centralizzato, ma può essere in varia misura anch'esso distribuito. Al fine di consentire lo sviluppo delle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tale regime consente a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione europea in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Si consente in tal modo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti. L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione europea in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT. Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, con le disposizioni del Capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari. Il Capo I, Sezione VII, del decreto-legge in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech. La sperimentazione FinTech è stata disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto crescita), il quale ha previsto la cosiddetta *regulatory sandbox*, ovvero un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e Ivass), potendo attualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio. Il Governo, nella relazione illustrativa, rileva che la prima applicazione delle regole che governano la *sandbox* ha evidenziato alcune rigidità

Il provvedimento è particolarmente tecnico, come abbiamo visto. Si evidenziano due scopi principali: il primo è quello di adeguare l'ordinamento italiano alla nuova disciplina del *pilot regime*, permettendo a quest'ultimo di confluire in una cornice civilistica certa, attraverso l'introduzione di una nuova modalità di emissione e circolazione di strumenti finanziari a regime distribuito. Il secondo scopo consente l'utilizzo della stessa cornice civilistica per l'emissione e la circolazione di strumenti non destinati alla negoziazione su una serie di attività, allineando l'Italia ad altri Stati europei, come Francia e Germania, solo per citarne due. Il decreto-legge permette l'emissione di strumenti finanziari digitali, e cioè in forma di rappresentazione di dati su un registro che utilizza la tecnologia DLT, quindi abbiamo una terza possibilità dopo i certificati cartacei e le registrazioni contabili. Il decreto-legge fissa dei requisiti affinché un registro che utilizza la tecnologia DLT possa supportare il nuovo regime di emissione e circolazione, misure che assicurano, ad esempio, la non riproducibilità del titolo e l'esclusività del possesso.

l'Italia è un Paese con tre principali caratteristiche, una delle quali è un elevato risparmio privato, che per anni è rimasto "parcheggiato" sui conti correnti, e i due anni di Covid hanno acuito questo aspetto. Negli scorsi anni, con un'inflazione sotto al 2 per cento, questo poteva essere considerato un potenziale inespresso; dal 2022 ad oggi, per contro, con un'inflazione che ha raggiunto la doppia cifra, la perdita di valore su risparmi equivale a decine di miliardi di euro. Il secondo aspetto è un tessuto imprenditoriale composto principalmente da piccole e medie imprese, la cui dimensione rende più complicati gli investimenti strutturali necessari per la digitalizzazione e per l'accesso alle opportunità finanziarie. Il terzo aspetto è proprio quello dell'introduzione della tecnologia DLT, della *blockchain*, dei registri distribuiti; determina l'aumento delle opportunità legando nativamente la caratteristica della disintermediazione a quella dello scambio di rappresentazioni di "scarsità",

Come Gruppo politico, il MoVimento 5 Stelle in questo contesto è sempre stato innovativo e ha sempre affermato con orgoglio la possibilità di guardare in avanti in questo percorso, e non siamo mai stati a guardare, anzi: proprio perché siamo nati in Rete, abbiamo sempre avuto ben presenti le opportunità che possono derivare dalla digitalizzazione del Paese.

sono entrati nella legislazione grazie al decreto-legge semplificazione nel 2019, dando riconoscibilità legale a questa nuova tecnologia. Sono numerose le azioni intraprese dai nostri parlamentari del Movimento 5 Stelle in tema di registri distribuiti

Tutto questo ha portato a tre risultati concreti: un accesso molto più semplice per le nostre piccole e medie imprese alle risorse finanziarie del nostro Paese, favorendo una loro ricapitalizzazione e determinando così nuovi e maggiori investimenti; proteggere il risparmio degli italiani, altro grande obiettivo, creando un'opportunità per l'impiego dell'economia reale di questo Paese e, come ultimo passaggio davvero importante, promuovere l'innovazione e la digitalizzazione stimolando la nascita e lo sviluppo del settore digitale che troppo spesso ha visto i nostri brillanti cervelli italiani fuggire all'estero, andare Oltralpe, e riscuotere grandissimo successo anche negli altri continenti. Venendo a questo provvedimento, tra gli aspetti positivi

Se vogliamo essere sinceri, in realtà, il codice civile italiano, essendo neutro, attualmente già consentiva soluzioni tecnologiche di qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto, fisico o digitale, ma ora finalmente abbiamo una norma che fuga tutti i dubbi, per cui c'è molta più chiarezza sul tema.

dato l'estremo tecnicismo, hanno bisogno di essere valutati (soprattutto le aziende hanno bisogno di conoscere l'argomento per poi adeguarsi e tutelarsi). L'altro aspetto è che il regolamento n. 858 del 2022, sui mercati digitali, è stato indicato dal Governo quale motivo d'urgenza e approvato con un decreto ed è al vaglio dei Paesi europei da molto tempo. La scelta di porre un testo particolarmente tecnico a ridosso dell'entrata in vigore del 23 marzo 2023 ha nei fatti eliminato completamente il dibattito su questo tema. Purtroppo, stiamo vedendo continuamente che il Governo Meloni opera rapidamente, nella notte, con urgenza, con decreti. Spesso la frettolosità di portare a compimento processi come questo rischia veramente di mettere in difficoltà

se infatti prima Consob e Bankitalia avevano competenza solo sui soggetti vigilati dalle società quotate e non intervenivano sulle piccole e medie imprese italiane e sulle regole del diritto societario, da

non c'è stato tempo di ragionare, né di fare uno scambio ben approfondito e quindi capire se è positivo o meno quanto spetta a questo decreto-legge. I poteri sanzionatori poi sono tanto estesi da non permettere di conoscere i limiti e le logiche dell'applicazione. Le autorità potranno irrogare sanzioni amministrative senza un preciso criterio oggettivo, introducendo il rischio di applicazione disomogenea e arbitraria delle varie norme.

e non è passato dalla valutazione esterna. Tale necessità avrebbe dovuto coinvolgere tutti gli *stakeholder* e soprattutto il mercato, perché si introduce un regime che si classifica come il più rigido d'Europa, creando una barriera all'ingresso per le piccole realtà, che a a questo punto incontreranno un ostacolo superiore nell'innovazione e nella digitalizzazione, nonostante le potenzialità del nostro ordinamento prima dell'entrata in vigore di questo decreto-legge; un ostacolo fatto dunque di burocrazia e costi,

Ringraziando per l'attenzione, Presidente, concludo dicendo che prendiamo atto del continuo modo di operare d'urgenza, senza ascoltare gli operatori italiani molto competenti che avrebbero potuto dare un grandissimo contributo in questa fase - e ce ne sono tanti che hanno queste capacità - ma non hanno potuto approfondire.

e va bene così, ma si continua nella stessa direzione.

che siamo qui oggi a esaminare intendono adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858 e mirano a introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech. In particolare, si inserisce una nuova definizione di strumento finanziario, includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia al registro distribuito. Vediamo quindi quali sono gli aspetti più importanti contenuti nel decreto-legge che sono stati esaminati in Commissione. L'articolo L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tra le definizioni più importanti abbiamo quella di forma digitale, con la quale si intende la circostanza che taluni strumenti finanziari esistano soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale, e poi quella delle tecnologie basate sui registri distribuiti, ossia tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile e verificabile da ciascun partecipante e non alterabile. il decreto-legge viene poi individuato l'emittente degli strumenti finanziari digitali e si individuano le infrastrutture di mercato DLT, nozione che comprende i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di negoziazione e regolamento. Negli articoli successivi, poi, si fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale e si individuano i pertinenti strumenti finanziari, lasciando fermi i limiti quantitativi previsti dalla normativa europea. Si prevedono l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, eseguiti attraverso scritturazioni, su un registro per la circolazione digitale, tenuto da un responsabile del registro, che può essere l'emittente, dal gestore di una delle infrastrutture di mercato, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale, individuandone le caratteristiche; si si chiarisce cioè che il registro deve assicurare l'integrità, l'autenticità e la non duplicabilità e consentire di identificare in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni; si deve consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate di accedere in qualsiasi momento. I registri devono prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati, consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere e garantire l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia. Vengono disciplinati anche gli effetti della scritturazione sul registro, con particolare riferimento alla legittimazione dell'uso degli strumenti finanziari e digitali e alle pretese di terzi. Le norme in esame chiariscono che la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente. Nel prosieguo si stabilisce che il principio della costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali è possibile unicamente mediante scritturazione nel registro; si individuano anche i soggetti che possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale; si dispone che possano essere iscritti le banche, le imprese di investimento e gli intermediari finanziari iscritti all'albo degli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia. Negli articoli finali vengono indicate le attività e i compiti da svolgere da parte della Consob ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei responsabili dei registri. Con l'articolo 30 si prevedono le sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative. Si introduce una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro. Si tratta quindi di un provvedimento molto tecnico e complesso, ben affrontato dal lavoro in Commissione, durante si è riusciti a far chiarezza su diversi aspetti che sicuramente potevano dare luogo a complicazioni. Ritengo pertanto che, grazie al lavoro svolto in Commissione,

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 maggio. L'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge per l'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, collegato alla manovra di finanza pubblica.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 Per quest'ultima è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. I tempi della discussione sono stati rimodulati in base a specifiche richieste dei Gruppi. La votazione a maggioranza assoluta non avrà luogo prima delle ore 16. Seguiranno le votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza, della giustizia amministrativa, della Corte dei Conti e della giustizia tributaria, per le quali è ugualmente necessaria la maggioranza assoluta. Le modalità di voto (a scrutinio elettronico su liste bloccate o mediante schede) potranno variare in relazione alle intese tra i Gruppi. Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti argomenti: dalla sede redigente, disegno di legge in materia di modifiche al codice della proprietà industriale e disegno di legge per l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati; deliberazioni sulla richiesta di procedura abbreviata per i disegni di legge in materia di circonvenzione di anziani e sulle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti; disegno di legge per l'avocazione delle indagini per delitti di violenza domestica o di genere. Giovedì 4 maggio si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*. La settimana dall'8 al 12 maggio sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà martedì 9 maggio, alle ore 11, per la discussione di ratifiche di accordi internazionali. La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo è convocata martedì 9 maggio, alle ore 13, per procedere alla sua costituzione. Lunedì 8 maggio, alle ore 11,30, si terrà nell'Aula del Senato una cerimonia celebrativa del 75° anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica.

«Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», collegato alla manovra di finanza pubblica. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

autonomie Calderoli Roberto Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il Documento di economia e finanza 2023 , presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, ha espressamente confermato la qualifica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 dell'Atto Senato 615. Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 23 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023. Inoltre, il provvedimento, composto di dieci articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento. Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

ringrazio, Presidente. Dicevo che l'obiettivo di questi due emendamenti è tutelare meglio i risparmiatori cosiddetti meno informati e meno esperti, soprattutto rispetto alle negoziazioni bilaterali del mercato *over the counter* (OTC), con scambi bilaterali in titoli, che sarà possibile effettuare più facilmente dopo la riforma che stiamo discutendo oggi. Questi emendamenti nascono da una semplice considerazione. Attualmente, quando un risparmiatore va a comprare un titolo di Stato tramite una banca, viene sottoposto a un insieme di

Si vanno a vedere le conoscenze e le esperienze in materia di investimenti, riguardo al tipo specifico di investimento e di prodotto, la situazione finanziaria del risparmiatore, compresa la capacità di sostenere certe perdite, e gli obiettivi di investimento del risparmiatore, compresa la tolleranza al rischio. La domanda che ci si deve porre è se non debbano essere poste in essere simili protezioni per le transazioni che verranno effettuate tramite il nuovo sistema di negoziazione di titoli che il decreto introduce. Alcune protezioni sono implicitamente applicabili in base al cosiddetto regolamento *pilot* dell'Unione europea, il 2022/858, in particolare agli articoli 4 e 5. Gli emendamenti proposti agli articoli 23 e 28 rafforzano queste protezioni soprattutto rispetto al mercato *over the counter* (OTC), che non è coperto dal regolamento europeo. Più specificatamente, l'emendamento 23.100 impone al responsabile di registro l'obbligo di verificare che i risparmiatori abbiano adeguate conoscenze relative ai tipi di investimento a cui dovrebbero avere accesso, in linea con gli *standard* della cosiddetta direttiva Markets in

con riferimento alle negoziazioni di strumenti finanziari digitali. In particolar modo, con questo emendamento, vorremmo avere anche maggiore certezza in merito all'identità del negoziatore,

quindi estendiamo sia alla Banca d'Italia, sia all'Ivass, sia alla Consob, una serie di deleghe per dare certezza alla negoziazione digitale.

Per creare simmetria rispetto alla proposta relativa alla lettera b) di cui al medesimo emendamento, si propone una lettera b-*bis)*: "*al comma 3, lettera a),* *le parole* «nei confronti dei» *sono sostituite dalle seguenti parole*: «con riguardo ai»".

di cui le criptoattività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle criptoattività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE va incontro al fenomeno della cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito. In estrema sintesi, un registro distribuito è un *database*, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione.

può essere in varia misura anch'esso distribuito. Al fine di consentire lo sviluppo delle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tale regime consente a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione europea in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni

L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione europea in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT. Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, con le disposizioni del capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari. Il capo I, sezione del decreto in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech. La sperimentazione Fintech è stata disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto crescita), il quale ha previsto la cosiddetta *regulatory sandbox*, ovvero un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e Ivass), potendo eventualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio. Il Governo, nella relazione illustrativa, rileva che la prima applicazione delle regole che governano la *sandbox* ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione, così anche le autorità di vigilanza hanno chiesto alcune modifiche. Con le norme in commento sono dunque introdotte misure di semplificazione volte a garantire la più ampia operatività della disciplina introdotta nel 2019. Per tale motivo, noi voteremo a favore del provvedimento in

è un provvedimento molto tecnico, come abbiamo potuto appurare dagli interventi che mi hanno preceduto, e riguarda un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi. Si dà in tal modo attuazione al regolamento europeo che prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate e si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza. Lo scopo dev'essere quello di consentire agli operatori FinTech di testare soluzioni innovative dal punto di vista digitale, in un costante dialogo con le autorità di vigilanza. Il FinTech non è solo l'utilizzo di uno strumento o di una nuova tecnologia, ma è un nuovo approccio alla finanza. La sfida, quindi, è definire un quadro di regole che consentnoa la crescita di un settore senza la cui espansione la finanza tradizionale italiana sarebbe destinata a restare indietro rispetto ad altri Paesi del mondo, che queste regole se le sono già date. Per queste semplici ragioni, quindi, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

disciplinandone la struttura tecnologica a registro distribuito (DLT), in cui consentire le negoziazioni elettroniche. Si tratta chiaramente di un passo in avanti sul fronte della semplificazione del processo di emissione, trasferimento e regolamentazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari. Il provvedimento in esame si è reso necessario in considerazione dell'applicazione, a partire dal 23 marzo 2023, del regolamento europeo n. 858 del 2022, che riconosce la possibilità di costituire piattaforme elettroniche di negoziazione di strumenti finanziari emessi in forma digitale in ambito europeo. di intermediazione finanziaria (TUF), introducendo un sistema di emissione e circolazione in forma digitale alternativo a quello cartolare e scritturale vigente, basato su un sistema di gestione unico e accentrato. Viene dunque introdotto un nuovo sistema di emissione e circolazione dematerializzato, grazie al quale le società italiane possono raccogliere capitali tramite emissioni e offerta di strumenti finanziari in forma elettronica tramite *token* (firma digitale). Il regolamento europeo limitava il nuovo regime sperimentale unicamente agli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati. La scelta del Governo è stata invece molto più radicale, poiché ha esteso la possibilità di ricorrere alla nuova struttura tecnologica a tutti gli strumenti finanziari, comprendendo sia quelli non destinati alla negoziazione sia quelli emessi da società non quotate. Scelte forse inopportune, visto il carattere sperimentale del nuovo ordinamento, sono la temporaneità della sperimentazione (tre anni) e la non conoscenza dei profili di rischio sottesi all'introduzione del nuovo regime di negoziazione. Il provvedimento consente di istituire plurime piattaforme elettroniche e particolari registri sincronizzati in rete con tecnologia DLT, dove trascrivere le negoziazioni certificando autenticità e validità giuridica. Queste potranno avvenire in qualunque momento della giornata, ossia ventiquattr'ore su ventiquattro, e con qualunque forma e sottoscrizione digitale. la scelta del Governo di prevedere una pluralità di piattaforme e registri digitali possa creare frammentazione nel nuovo mercato digitale, con conseguenti implicazioni negative in termini di concorrenzialità, efficienza, stabilità, sicurezza e legalità. È noto infatti che la tecnologia *blockchain* non è certamente immune da rischi di *cyber security*,

gli operatori e i soggetti responsabili della rete digitale e delle negoziazioni. Importante sarà l'attività delle autorità di vigilanza che dovranno garantire sicurezza e legalità di funzionamento, intervenendo e prevenendo frodi e manipolazioni solo parzialmente attenuati con la regolamentazione *sandbox* prevista dal decreto-legge. Il decreto-legge in esame presenta inoltre criticità anche con riferimento ai requisiti di funzionamento di tali registri e degli operatori autorizzati alla loro gestione e a curarne le trascrizioni. A differenza degli strumenti finanziari di società quotate che seguono il regolamento europeo del sistema DLT, il decreto prevede per gli strumenti finanziari non regolamentati che il registro possa essere tenuto, oltre che da operatori istituzionali - banche, imprese di investimento, intermediari finanziari - anche da soggetti che non esercitano abitualmente l'attività finanziaria, quindi soggetti non professionali e non operanti nel settore finanziario. Tale discutibile decisione da parte del Governo riteniamo che possa impedire alle autorità di vigilanza di essere informate e di intervenire tempestivamente e preventivamente in caso di anomalie e di irregolarità nelle negoziazioni. Il procedimento previsto per iscriversi poi nell'elenco degli operatori responsabili dei registri di negoziazione digitale non contempla requisiti specifici e stringenti di professionalità, non sono garantiti pertanto *standard* qualitativi simili a quelli richiesti dalla direttiva Mifid, soprattutto in tema di antiriciclaggio e adeguata verifica, nonché di valutazione dei rischi sui risparmiatori generalmente non educati finanziariamente, così come non si prevede alcuna valutazione sulla conoscenza stessa della tecnologia DLT. Sempre in tema di sicurezza, non si prevede un particolare titolo idoneo a dare certezza alla negoziazione, così come non si garantisce l'identità digitale, soprattutto con riferimento ai titoli di partecipazione al capitale. Ciò non mancherà di favorire raggiri e controversie, che potranno limitare la competitività del sistema e la sua capacità di attrarre investimenti. Ravvisiamo inoltre rischi sull'efficacia dei controlli antiriciclaggio, soprattutto per la scelta del Governo di abilitare alla negoziazione anche operatori non intermediari finanziari. Questa per noi è una vera assurdità. Il nuovo ordinamento giuridico, così come proposto, rischia quindi di vanificare la buona riuscita della sperimentazione proprio per il venir meno dei requisiti fondamentali in tema di trasparenza, sicurezza e legalità delle negoziazioni e di tutela del risparmio. del risparmio. Il provvedimento in discussione presenta ancora diverse approssimazioni, lacune e criticità nei confronti delle quali il MoVimento 5 Stelle ha presentato diversi emendamenti che il Governo ha ritenuto in buona parte di non accogliere, Il MoVimento 5 Stelle ha nel suo DNA la condivisione dell'innovazione tecnologica come strumento per semplificare e migliorare la vita dei cittadini e delle imprese, aumentandone conoscenza, consapevolezza e potenzialità. Siamo consapevoli che l'innovazione tecnologica richiamata dal decreto possa essere un volano formidabile anche applicata alla finanza, a patto però che questa generi benefici per l'economia reale, rafforzando i canali alternativi di afflusso di capitali alle piccole e medie imprese. Siamo e resteremo contrari, invece, alla sottomissione della tecnofinanza alle sole ragioni dell'economia di carta e della speculazione. Per questo stigmatizziamo tutti i passaggi del decreto-legge in cui il Governo estende la sperimentazione delle tecnologie al registro condiviso anche a strumenti finanziari non negoziati, getta le premesse per la proliferazione di piattaforme non interoperabili, consente di affidare il controllo sui registri anche a soggetti non professionali dal punto di vista finanziario, non garantisce l'identità digitale degli investitori e quindi non assicura legalità e trasparenza. In conclusione, Presidente, riteniamo che il provvedimento sia ancora migliorabile, soprattutto con riferimento ai presidi antiriciclaggio e di sicurezza a tutela del risparmio e dei risparmiatori. Il Governo avrebbe dovuto quindi dedicare maggior riflessione, tempo e attenzione alla fase consultiva, in considerazione delle novità, delle innovazioni e dei rischi sottesi che potrebbero compromettere le grandi opportunità del nuovo ordinamento. Anche in questo Anche in questo caso, quindi, il Governo non si è dimostrato pronto. Di fronte alle vostre incapacità, sarebbe stato forse meglio limitare il provvedimento a recepire semplicemente il regolamento europeo, senza forzare fughe in avanti che rischiano di minare la fiducia degli investitori e le attese delle imprese. Per tutte queste ragioni esprimo, a nome del MoVimento 5 Stelle, il voto di astensione, nella speranza che il provvedimento in esame possa ancora essere migliorato in seconda lettura, anche a seguito di un approfondito dibattito istituzionale e politico. *(Applausi)*.

difficile da affrontare dal punto di vista normativo, perché ci sono molti aspetti tecnici, però nella vita comune dei cittadini sta diventando la norma (basti pensare ai sistemi di pagamento). Con questo intervento, com'è già stato detto, si attua il regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. In buona sostanza, si disciplina l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari in forma digitale. Siccome è un argomento oggettivamente complesso, in Commissione finanze, con i colleghi di maggioranza e opposizione - che colgo l'occasione per ringraziare per la pazienza e la professionalità con cui hanno seguito questa spigolosa materia - abbiamo organizzato un ciclo di audizioni, perché mai come in questo caso il principio "conoscere per deliberare" è sacrosanto, proprio per la complessità della materia. Abbiamo sentito quindi Consob, Banca d'Italia e associazioni di consumatori; abbiamo acquisito memorie da diversi soggetti proprio per arrivare a comprendere rischi e opportunità di questo intervento, visto che si tratta di un intervento di grande rilevanza,

velocità che questa nuova piattaforma - chiamiamola così - imprime al sistema finanziario. Questa è la grande opportunità. I rischi,

È stato detto che è un'operazione di carattere sperimentale - questo è un punto chiave - e proprio perché è sperimentale si fa un grande salto in avanti, però con buon senso. La Commissione e i commissari hanno previsto che ci sia da parte

creino sviluppo. Non ci possiamo permettere di non essere al passo con i Paesi più veloci in questo campo. *(Applausi)*.

su questo, quindi, ma vorrei affrontare una questione più generale e più importante per il voto sul provvedimento. Al di là dei tecnicismi (è un decreto molto tecnico),

da anni gli scambi avvengono su mercati organizzati in via telematica. Il decreto-legge che attua il regolamento dell'Unione europea sul DLT

queste tecnologie sono state introdotte per la negoziazione di criptovalute. Il punto principale, com'è stato ribadito in diversi interventi, è che le negoziazioni d'ora in poi potranno avvenire ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni alla settimana,

decreto-legge in esame va oltre quello che era strettamente necessario per implementare la direttiva dell'Unione europea, ad esempio estendendo

c'è una riduzione potenziale della segmentazione dei mercati nazionali, con accesso anche a piattaforme di una più ampia platea di operatori. Inoltre, c'è la necessità di adeguarsi a quello che fanno gli altri Paesi, anche se siamo andati molto oltre. però di un cambiamento radicale nel funzionamento dei mercati finanziari ed è innegabile che esistano rischi. La Banca d'Italia, infatti, in sede di audizione, ha parlato proprio di innegabili rischi. Al di là degli aspetti più tecnici che riguardano tali rischi, ci si deve fare una domanda. Anni fa, il premio Nobel dell'economia James Tobin disse che sarebbe stato opportuno mettere un po' di sabbia negli ingranaggi dei mercati finanziari, che già operavano a una velocità molto elevata. Tobin parlava in un contesto diverso e chiedeva di introdurre una tassazione sulle transazioni finanziarie, ma l'idea generale è la seguente: attenzione, perché i mercati finanziari che funzionano vanno bene, ma mercati finanziari che si muovono un po' troppo rapidamente possono creare problemi e causare crisi, ondate di panico e cose di questo genere. Un po' di sabbia negli ingranaggi quindi forse non è una cattiva idea. Questo provvedimento non solo non mette sabbia negli ingranaggi, ma vi aggiunge olio per far funzionare tutto molto più rapidamente.

Mi meraviglio del fatto che sia stata presa in maniera abbastanza leggera l'idea che l'innovazione finanziaria vada bene in ogni caso e quindi mettiamo ulteriore olio nel funzionamento dei mercati finanziari. un sistema introdotto in via sperimentale, pilota, ma per diversi anni. In ogni caso, il fatto che sia stato introdotto come progetto pilota suggerisce che ci sono diverse perplessità. A fronte dei potenziali vantaggi che ho citato, ma anche dei rischi esistenti e della perplessità di fronte a passi che potrebbero favorire un'ulteriore iperfinanziarizzazione dell'economia, il Gruppo Partito Democratico ha deciso di astenersi su questo provvedimento. *(Applausi)*.

su uno strumento così complesso da condividere, anche per chi come noi è stato in Commissione, abbiamo messo massima prudenza e grande attenzione. È normale che nel campo degli algoritmi e dell'innovazione digitale il nostro Paese dovesse fare i conti con il tempo (lo dico anche ai colleghi che dicono che il nostro Governo ha innovato tanto). Paghiamo qualche ritardo rispetto all'applicazione, cioè alla data

assicurativo e finanziario, quindi i risparmi. È importante la velocità con cui il nostro Paese è in grado di intercettare, su un mercato finanziario che evolve velocemente, i risparmi italiani, europei e internazionali. Questo

collaborazione con i principali istituti universitari di questo Paese, per far sì che la sperimentazione italiana (cioè l'ulteriore innovazione) possa essere foriera di un confronto internazionale e porre l'Italia, su uno strumento così

Concordo con alcuni rilievi di prudenza che vengono posti dalla minoranza o da una sua parte.

va oltre questo regolamento e sperimenterà qualcosa in più, per offrirlo al confronto con il mercato internazionale (non siamo chiusi). Per una volta superiamo quell'Europa che

Come precedentemente comunicato, l'informativa del ministro Fitto è prevista per le ore 14. La seduta è sospesa.

dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rimettendo in ordine gli aspetti più salienti e importanti dell'impegno del nostro Governo, che, come noto, è partito il 23 ottobre 2022.

saranno poi oggetto di un approfondimento dettagliato, nel mese di maggio, quando sarà presentata la relazione semestrale, che costituirà una fotografia molto ampia e molto più completa di quanto non possa essere un'informativa. Partirò da un dato, che è stato oggetto di considerazioni in più circostanze, sulla scelta iniziale che il presidente del Consiglio Meloni ha messo in campo, allorquando ha individuato, nella composizione delle deleghe, la necessità - oserei dire l'obbligo - di mettere insieme le deleghe per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la costituzione di un Ministero *ad hoc* per affrontare la dimensione del Piano,

abbastanza preoccupante il quadro di riferimento, che fa emergere un 34 per cento di spesa, a fronte di 126 miliardi di euro, dopo non sei anni, ma nove, visto che siamo a febbraio. Questo, per la parte europea, è ancor più preoccupante, visto che eravamo nella fase conclusiva della rendicontazione della programmazione 2014-2020, che sarà appunto quella del 31 dicembre di quest'anno. È evidente che, in questo contesto, il Governo ha iniziato il suo lavoro per quanto riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza sulla prima grande questione, che era quella del raggiungimento, poco dopo due mesi dall'atto dell'insediamento, dei 55 obiettivi utili per poter fare richiesta - e quindi ottenere - per il raggiungimento della terza rata, di 19 miliardi di euro. Al momento dell'insediamento il Governo ha trovato 25 obiettivi raggiunti. Sugli altri 30, nei due mesi successivi, c'è stato un lavoro molto intenso, con i Ministeri e con tutte le amministrazioni interessate all'attuazione e all'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per trovare il modo di raggiungere questo risultato. Il risultato è stato raggiunto al 31 dicembre: i 55 obiettivi sono stati inviati alla Commissione europea ed è iniziato un momento di confronto, così come regolarmente viene fatto con tutti i Governi nazionali che hanno la possibilità di gestire questi programmi, nel senso che il cosiddetto *assessment* riguarda una verifica della correttezza del raggiungimento degli obiettivi. Questa fase si è sviluppata nei mesi successivi e, nella fase finale, abbiamo immaginato anche, d'intesa con la Commissione europea, per alcuni obiettivi sui quali da qui a breve tornerò in modo specifico, di prendere un mese di tempo in più, per poter definire meglio, nel rapporto con la Commissione, il superamento di alcuni ostacoli e di alcune problematiche, per risolvere alcune questioni. I diversi obiettivi, su cui è stata fatta una verifica, sono sostanzialmente raggiunti. Su tre in modo particolare si è concentrata l'attenzione della Commissione europea, per una diversa valutazione sui diversi obiettivi e sul loro raggiungimento. Il primo è quello ormai noto alle cronache e relativo ai piani urbani integrati, cioè all'inserimento del piano urbano di Firenze con lo stadio «Artemio Franchi» e quello relativo al piano urbano di Venezia con il «Bosco dello sport», due interventi che sono stati oggetto di un confronto con la Commissione europea. È noto che ho avuto direttamente degli incontri con i sindaci di Firenze e di Venezia,

del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, questi due interventi erano stati inseriti all'interno dei rispettivi piani urbani integrati e del decreto complessivo di approvazione dei citati piani. Vorrei altresì sottolineare il fatto che anche nella relazione semestrale in Parlamento i piani urbani integrati, così come definiti dal provvedimento, erano stati considerati un obiettivo raggiunto. Sulla base di questo lavoro si è aperto un confronto con la Commissione europea, che si è concluso con la valutazione negativa da parte della Commissione stessa sulla possibilità di considerare questi due interventi finanziabili all'interno del PNRR con risorse europee. In queste ore il Governo sta predisponendo i documenti per affrontare e risolvere la questione e quindi superare questa difficoltà, salvo restando che

inviato e concluso il percorso al Consiglio di Stato il 25 ottobre 2022, sono state definite le linee guida. Si è aperto un confronto con la Commissione europea rispetto al quadro rafforzato e regolatorio, soprattutto relativamente al coinvolgimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Si è svolto un lavoro di confronto con la Commissione e, in data 21 aprile 2023, è stato approvato il nuovo decreto ministeriale, d'intesa con il ministro Salvini, che ha superato le osservazioni e che noi riteniamo

Con un bando pubblicato il 30 giugno 2022, sul quale la Commissione europea ha sollevato una serie di questioni relative all'inammissibilità di alcuni interventi, abbiamo definito un percorso con la Commissione stessa in base al quale il superamento - e quindi la non finanziabilità - di alcuni interventi sarà recuperato con la pubblicazione di un nuovo bando concordato. Per quanto riguarda la rata del 31 dicembre 2022, si proseguirà in queste ore con l'invio di ulteriore documentazione in un confronto confronto costante e propositivo con la Commissione europea per raggiungere quest'obiettivo che, com'è evidente, nelle prossime ore dovrà trovare una soluzione, anche perché si completa il mese individuato come ulteriore proroga.

132 *milestone*, 19 *target*, dai quali emergono in modo molto chiaro alcune criticità relative al ritardo della fase di avvio degli interventi, ai tempi di presentazione ed attuazione dei progetti, alla parcellizzazione degli interventi rispetto agli obiettivi e alla capacità amministrativa dei soggetti attuatori e, infine, a un dato altrettanto importante e rilevante, l'aumento del costo delle materie prime, che, com'è evidente, incide non poco su un programma che complessivamente arriva a 110 miliardi di euro in riferimento al numero delle opere pubbliche. È evidente che questo rappresenta una dimensione che, se riportata sulla questione dell'aumento del costo delle materie prime, è certamente uno dei temi che vanno affrontati con la massima attenzione. In questo contesto si è inserita - perché è stata oggetto anche del dibattito a livello nazionale - la relazione della Corte dei conti,

recentemente è stato varato dal Parlamento, nel quale il Governo ha affrontato complessivamente il tema della *governance*,sia relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia - per le ragioni che ho detto all'inizio del mio intervento - in relazione alla politica di coesione, insieme a una serie di norme e di interventi interventi sul fronte della semplificazione. Sono emersi in più circostanze critiche e rilievi sul fatto che il Governo, avendo messo mano alla *governance*, si è assunto la responsabilità di compiere un'azione dilatoria che ha portato a ritardi e perdite di tempo. A me piace però su questo rimanere nel merito delle questioni, perché il Governo è stato molto attento a evitare che ciò accadesse. Non è un caso che il decreto non abbia trovato una sua attuazione

l'eventuale nomina di qualsiasi figura dirigenziale potrà essere completata solamente quando le due figure dirigenziali - quella che attualmente c'è e quella che dovesse eventualmente subentrare - troveranno un punto di coincidenza. Quindi non c'è semplicemente non ci può essere per ragioni oggettive quello che da più parti ascolto come criticità, per il fatto che la fase di attuazione della nuova *governance* non c'è ancora stata e - lo ripeto - la firma odierna del DPCM va in questa direzione.

il Governo ha proposto e che il Parlamento ha convertito in legge nei giorni scorsi. Mi riferisco in modo particolare ad alcuni elementi che sono emersi anche dal confronto

amministrativa dei soggetti attuatori trovi una risposta importante nel decreto-legge già varato e un altro pezzo di risposta altrettanto importante, richiesto da questi interlocutori, all'interno però del decreto n. 44, in via di conversione, il cosiddetto decreto pubblica amministrazione,

caso, parlare delle unità di missione e del loro smantellamento non corrisponde alla realtà dei fatti perché, alla luce del suggerimento e dell'indicazione della Corte dei conti e della richiesta dei sindacati in sede di cabina di regia da dove si chiedeva con decisione il rafforzamento delle unità di missione - il Governo ha predisposto la stabilizzazione del personale a tempo determinato per rafforzare queste figure e, soprattutto, per consolidare nella loro azione le unità di missione presso i singoli Ministeri. Questo è un altro elemento centrale che ha rappresentato una scelta da parte del Governo. In questo contesto, ci avviamo alla fase di confronto questioni più importanti, collegate alla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, legata sia ai temi del Repower, quindi alle decisioni assunte, con l'approvazione del regolamento Repower, da parte della Commissione europea, sia soprattutto ad un'altra questione fondamentale, quella sulla quale lavoriamo in corsa, che, proprio alla luce dell'esperienza di quanto poc'anzi citavo relativa al raggiungimento degli obiettivi e alle criticità al 31 dicembre del 2022, porta il Governo a invertire il meccanismo e ad affrontare per tempo le questioni collegate alle criticità degli obiettivi al 30 giugno, per poter avere con la Commissione europea non un confronto nella fase successiva

è evidente che stiamo lavorando su alcuni aspetti collegati al raggiungimento dei 27 obiettivi e lo vogliamo fare soprattutto in riferimento ad alcuni elementi che vorrei citare puntualmente. Farò tre esempi rispetto agli obiettivi obiettivi del 30 giugno, perché sono calzanti e possono spiegare bene, cambiando il contesto e aumentando le criticità, l'esigenza di intervenire preventivamente non per rischiare di perdere gli interventi, ma per correggere alcuni obiettivi intermedi, con la finalità di mantenere il risultato e il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia il mantenimento della spesa di quel determinato obiettivo. obiettivo. Mi riferisco in modo particolare al piano per gli asili nido e alle scuole dell'infanzia, nonché ai servizi di educazione per la prima infanzia, per i quali ci sono innanzi tutto due differenze, che ci accompagneranno anche nei prossimi mesi per avere un quadro chiaro, tra i cosiddetti progetti in essere, i progetti esistenti prima dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che sono stati inseriti al suo interno e i nuovi progetti. È una differenza non di poco conto, che vorrei sottolineare, perché rappresenta e rappresenterà, anche dal punto di vista dell'attuazione, un elemento di riflessione molto importante, al quale aggiungo un altro elemento importante, che è una sorta di ricostruzione di questo aspetto, che serve a capire anche le criticità e il senso delle soluzioni che vogliamo immaginare nel confronto con la Commissione europea. Il 22 marzo 2021 e il 2 dicembre del 2021 sono stati individuati, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli interventi dei quali ci occupiamo, ed è evidente che il valore complessivo di 4,6 miliardi di euro, in questi tempi che ho individuato, ha portato ad accumulare un ritardo complessivo che rischia di mettere in discussione la possibilità per tutti gli interventi di avere affidati i lavori al giugno 2023. Cosa fa il Governo su questo? si confronta con la Commissione europea (verso l'alto) e fa lo stesso con l'ANCI (verso il basso), perché è evidente che non tutti gli interventi sono nella stessa situazione.

Un secondo analogo esempio che vorrei fare, abbastanza semplice e di facile comprensione, è relativo alla sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale: semplicemente il numero delle domande è stato inferiore alla disponibilità finanziaria. Cosa si fa in questo caso? Di chi è la colpa? Ci si siede a un tavolo con la Commissione europea e si rimodula l'obiettivo. Non penso si possa dire che

complessivi di progetto e soprattutto di risoluzione di alcuni contenziosi che sono al suo interno, difficilmente potrebbe raggiungere il risultato. Ho fatto questi tre esempi per dimostrare come tre questioni che vengono rappresentate all'esterno come esempi di una responsabilità drammatica sono e devono essere oggetto di una revisione costante in corso d'opera, perché l'intero programma - l'ho già detto in altre circostanze e lo voglio ribadire - dev'essere oggetto di una revisione costante per avere la capacità, modificando alcuni degli obiettivi in corsa, di raggiungere l'obiettivo finale. Cosa diversa è, invece, l'elemento di riferimento rispetto al completamento dei progetti al giugno del 2026, sul quale tornerò successivamente. È altrettanto importante ribadire che questo lavoro relativamente agli obiettivi di giugno per noi

l'obiettivo e la prospettiva di dicembre o di giugno, ma deve inevitabilmente porsi come strategia quella del giugno del 2026, per poter operare, così come in fase di correzione in corsa in pochi giorni al 31 dicembre e con un anticipo invece di oltre due mesi in questa fase al 30 giugno, su tutti gli altri obiettivi che ci accompagneranno al giugno del 2026, per avere adesso il quadro di riferimento e per immaginare ora ora modifiche concordate con la Commissione europea che sono determinate da diversi fattori: quelli ai quali ho fatto riferimento prima, quello collegato all'aumento del costo delle materie prime e quello più semplicemente collegato al cambio di obiettivi strategici che abbiamo di fronte. Come abbiamo ricordato in più circostanze - su questo penso che tutti possiamo essere assolutamente d'accordo - il Piano nazionale di ripresa e resilienza (dico una cosa ovvia, ma la voglio sottolineare) è stato immaginato prima dell'invasione dell'Ucraina

immaginare un riferimento allo strumento di modifica principale, cioè il regolamento Repower EU, che la Commissione europea ha approvato nella fase di verifica del cambio degli obiettivi e delle strategie dopo lo scoppio della guerra. La Commissione ha quindi immaginato, con l'approvazione del Repower, un sistema per il quale i singoli Paesi membri possano preparare il loro programma, che diventerà un capitolo aggiuntivo, quindi andrà a modificare e a implementare il Piano nazionale di ripresa e resilienza per poter raggiungere alcuni degli obiettivi fondamentali che si trovano degli obiettivi del Repower, che quindi possono essere oggetto di scelta da parte dei singoli Paesi membri e che accompagneranno la fase di rimodulazione. In questo contesto, è molto importante ricordare la dimensione finanziaria del Repower: il nostro Paese otterrebbe

realizzati. Penso sia indispensabile parlarne ora o vogliamo trovarci, ad ogni scadenza di obiettivo, con le difficoltà che stiamo affrontando per la rata del 31 dicembre 2022? Penso che sia indispensabile ragionare immediatamente per capire quali obiettivi correggere e quali di questi interventi non saranno raggiunti. Per far questo il Governo ha messo in campo un'azione che parte da una scelta contenuta nel decreto-legge e che, nella sua fase di attuazione, trova un momento molto importante di confronto: lo dico perché sin dal primo momento abbiamo scelto di avere la cabina di regia come luogo di confronto costante. Qui non voglio fare polemica con nessuno, ma prendo atto del fatto che c'è una visione diversa rispetto al ruolo della cabina di regia.

scelto di non tagliare il cavo del partenariato, ma di rafforzarlo, se è vero com'è vero che, per esempio, proprio sul Repower abbiamo fatto una serie di incontri di cabine di regia con i Comuni, le Regioni e le Province per chiedere loro di avanzare proposte. Abbiamo ottenuto un incontro a Palazzo Chigi - lo ha ottenuto il presidente Meloni - alla presenza di tutti i Ministri interessati con gli amministratori delle principali aziende di Stato (ENI, Enel, Snam e Terna) per poter avere con loro un confronto e recepire proposte concrete su tutti gli obiettivi da raggiungere all'interno del Repower, così come indicato dalla Commissione europea.

il grande tavolo di tutti i partecipanti; abbiamo deciso invece di dedicare un pomeriggio in cabina di regia, tenendo diversi incontri settoriali con tutte le organizzazioni di categoria, per avere da ognuna di loro

con tutti i soggetti che possono dare un contributo in questa direzione. Il tema del capitolo Repower è molto rilevante, non solamente

strategica rispetto a questa grande opportunità. Al tempo stesso, troverà al suo interno un obiettivo fondamentale, quello di poter immaginare forme di incentivi per ridurre i consumi ed efficientare le soluzioni per famiglie e imprese. Anche questo è un tema molto importante che può rappresentare uno degli elementi di novità assoluta in questa direzione. Su questi aspetti

hanno le caratteristiche oggi di rischiare di non essere realizzati entro il mese di giugno del 2026. Dobbiamo dirci con chiarezza - cosa che abbiamo già fatto ma penso che sia opportuno sottolinearlo - che il lavoro che il Governo sta mettendo in campo non è casuale. non è casuale. Con tutti i Ministeri e con tutti coloro i quali sono al lavoro nella fase di attuazione, stiamo verificando verificando il livello di avanzamento, perché non manca molto al momento del completamento del programma: siamo a tre anni e due mesi dalla data entro la quale tutto l'intero programma dev'essere complessivamente realizzato con gli interventi finali. È evidente che oggi oggi abbiamo la possibilità di comprendere quali di questi interventi non possono essere realizzati a quella data e capire come rimodularli, mentre tra tra qualche mese o tra un anno questo lavoro non potrà più essere fatto e rischieremo di trovarci in una situazione paradossale nella quale, non completando l'intervento, ci troveremo in difficoltà e in difetto rispetto al finanziamento europeo e all'impossibilità di fare cambiamenti perché l'intervento avrà una fase avanzata e quindi rischierà di aprire un grandissimo contenzioso. Ragionare oggi,

con il completamento della valutazione di questi interventi, che sarà anch'esso oggetto di un confronto con il Parlamento: non è che il Governo modificherà il Piano nazionale di ripresa e resilienza senza aprire un confronto in tutte le direzioni e con il Parlamento - ci mancherebbe altro - ma lo farà soprattutto sulla base di un lavoro con i singoli Ministeri e con tutti gli enti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo voglio dire in Parlamento in modo molto chiaro: evidentemente, di fronte a questo, ci sono enti attuatori che dovranno garantire, assumendosene la responsabilità, la realizzazione dell'intervento entro giugno 2026. A fronte di detta garanzia pubblica e ufficiale, il Governo si sentirà molto più tranquillo ed eviterà di trovarsi nella condizione, da qui a qualche tempo, di immaginare che tutto l'eventuale rischio di mancata realizzazione degli interventi venga scaricato sul Governo.

attuatrici e avremo un quadro chiaro, potremo portare in Parlamento questa dimensione e, com'è evidente, ci ritroveremo - da qui a breve, peraltro - con la prima relazione semestrale del nostro Governo sul Piano nazionale sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Infatti, tra fine aprile e i primi di maggio scadrà il termine dei sei mesi e quindi nel mese di maggio il Governo presenterà una relazione semestrale con una una valutazione molto complessiva e molto documentata, che avrà al suo interno tutta una serie di aspetti specifici che saranno una fotografia dettagliata della singola situazione all'interno degli obiettivi e delle misure, quindi complessivamente una base per costruire una dinamica una dinamica di confronto anche rispetto alle criticità esistenti. Vorrei concludere con una considerazione assolutamente positiva.

le difficoltà e i problemi esistenti, non per aprire un dibattito sui problemi - voglio essere molto chiaro su questo - ma per immaginare le soluzioni nei tempi previsti dai regolamenti europei. È questo l'approccio che il Governo vuole mettere in campo, perché è fin troppo evidente l'obiettivo che abbiamo: raggiungere il risultato della spesa dell'intero programma. È altrettanto evidente che, nel voler raggiungere quest'obiettivo, è necessario oserei dire fondamentale - in questo confronto con la Commissione europea e con l'intero sistema delle autonomie locali e degli enti attuatori, trovare e correggere oggi le criticità, per poter avere domani la soluzione dei problemi e un rapido avanzamento della spesa e soprattutto del percorso di riforme che accompagna l'intero Piano nazionale di ripresa e resilienza. da più parti viene richiamato un appello del presidente della Repubblica Mattarella, che il Governo fa suo; lo fa suo con l'obiettivo non solo ma con la consapevolezza e la convinzione di volerlo attuare, perché la cosa più complessa è l'attuazione di questo programma. Il Governo lo vuole fare in modo positivo e soprattutto con la consapevolezza della rilevanza della partita che ha di fronte; lo vuole fare anche spiegando che

a quello che più volte è stato indicato come un ruolo centrale, quello del Parlamento (e ci mancherebbe altro). Ho avuto modo di partecipare diverse volte ai dibattiti in Commissione e in Parlamento. Il Governo non si chiamerà

ma anche laddove il Parlamento, nelle Commissioni e in Aula, dovesse ritenere necessario un approfondimento di merito sulla fase di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, c'è la piena disponibilità del Governo a farlo nel merito, è il merito della questione quello che ci interessa e non solamente la contrapposizione. L'augurio e l'auspicio è che si individuino il clima e l'approccio corretto per dare al nostro Paese l'attuazione piena di questo importante strumento. l'obiettivo del Governo e su questo noi lavoreremo con serietà e responsabilità. Signor Presidente, signor Ministro, sarà la collega Gelmini a indicare, per il nostro Gruppo, una valutazione complessiva sulla sua informativa, della quale la ringraziamo. Aggiungo che, nel momento in cui il Governo è impegnato a spendere dei soldi europei per tutti gli italiani, anche chi, come noi, sta all'opposizione ovviamente fa il tifo per voi e lavora in una logica di dialogo costruttivo. Con questo spirito, signor Presidente, mi permetta di rivolgere al Ministro un appello relativo a un punto specifico, perché penso che tutti noi senatori siamo comunque legati al nostro territorio. È inutile fare gli interventi sempre e soltanto sulla crisi nel mondo e non parlare del proprio collegio. Io parlo di Firenze, perché aver introdotto lo stadio di Firenze tra le opere da finanziare con il PNRR è stato un errore. *(Applausi)*. L'ho detto un anno fa e lo ribadisco oggi. I 55 milioni di euro dei fondi europei che l'Europa ci ha negato non nascono da una visione cattiva dell'Europa, che non ama l'Italia o che fa uno sfregio a Firenze, ma nascono da un nostro errore in partenza. È un *assist* per gli euroscettici (guardate la stampa internazionale cosa ha detto di questa operazione) ed è un autogol per l'Italia.

è stato vincolato persino sulle curve. Ora, chi conosce Firenze mi deve trovare un solo esperto di arte, di turismo e di cultura che venga a Firenze per vedere la curva Ferrovia. A Firenze si può venire per vari motivi: si può venire per le opere d'arte più importanti, si può venire persino per le scale elicoidali del Nervi (anche se allo stadio è più complicato che ciò avvenga). Ma che si venga a vedere la curva Ferrovia! Vengono i tifosi avversari in curva Ferrovia, come sanno alcuni ex ultrà che sono presenti in questo Parlamento. Allora vengo alla proposta, e ho chiuso. C'è un uovo di Colombo potenziale e noi siamo propositivi. Signor Presidente e, per suo tramite, signor Ministro, noi abbiamo 55 milioni dei fondi europei. Il sindaco di Firenze legittimamente eletto (non voi, non io, nessun altro) scelga tra le case popolari, le scuole e i parchi su cosa investire questi 55 milioni. Scelgano il sindaco e l'amministrazione, non noi. I 90 milioni che il Ministero della cultura (Mic) ha messo sul fondo complementare vadano alle opere culturali che servono a Firenze: alla Biblioteca nazionale, all'Opificio delle pietre dure, agli Uffizi, che sono rilevanti almeno quanto la curva Ferrovia. Si permetta, tutti insieme, di eliminare il vincolo, non sulle scale elicoidali, non sulla tribuna, non sulla torre di Maratona, ma solo sulle curve, così che lo stadio - come accade in tutto il mondo - lo facciano i privati coi soldi dei privati. A quel punto, salviamo i 55 milioni del PNRR, salviamo i 90 milioni del Ministero della cultura, che saranno destinati finalmente agli interventi che servono a Firenze, e non ci facciamo ridere dietro da tutta Europa. Mi sembra una proposta di buon senso.

Signor Presidente, oggi in Aula abbiamo ascoltato con molto interesse l'informativa del ministro Raffaele Fitto, che ringrazio, sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Faccio una premessa. Il PNRR è stato approvato due anni fa, nel 2021. Le cinque missioni e i 55 obiettivi sono stati concepiti in quel momento, in un periodo storico completamente diverso rispetto a quello attuale. Non c'erano come ha ricordato anche il Ministro prima - la guerra in Ucraina, la crisi energetica, l'inflazione a due cifre, i rincari dei materiali e tantissime altre situazioni che oggi sono completamente diverse rispetto a prima. Oggi - come ha evidenziato lei, signor Ministro - c'è la necessità di rimodulare il Piano e per questo motivo questo Governo si è mosso concretamente, avviando un negoziato con le istituzioni europee proprio allo scopo di utilizzare al meglio tutte le risorse. Sono queste le ragioni che ci hanno spinto a sostenere e approvare la scorsa settimana, con l'ultimo passaggio alla Camera, il decreto di attuazione del PNRR, con l'obiettivo di snellire le procedure tecniche e semplificare il processo. Grazie a questo Governo, dunque, è stata ripensata la *governance* del Piano, per renderla più efficace ed efficiente. Oggi, per il bene dell'Italia e degli italiani, è essenziale - secondo noi -rivedere i progetti e spendere bene le risorse del PNRR. Questa partita è di destra o di sinistra? La domanda, chiaramente, è retorica e la risposta è altrettanto scontata. È una partita di tutti gli italiani, di tutti noi. E i cittadini vogliono sapere se e come vengono spesi i soldi. Quindi, devono essere spesi bene. Le criticità espresse oggi dall'Europa al PNRR non sono rivolte a questo Governo, ma sono critiche oggettive. Adesso, però, bisogna affrontare il tema della capacità di progettazione e di spesa degli enti locali e della pubblica amministrazione; fattori che, tra l'altro, lo stesso Governo Draghi aveva sottolineato nella NADEF che presentò lo scorso anno. Solo attraverso competenze adeguate possiamo garantire, a cittadini e imprese, servizi pubblici di maggiore qualità. Ecco perché oggi è centrale sciogliere questo nodo, ovvero mettere gli enti attuatori del PNRR nelle condizioni di fare bene il proprio lavoro, in sinergia chiaramente con le istituzioni centrali. La maggior parte dei progetti del PNRR è in capo ai Comuni. Parliamo del 65 per cento dei progetti presentati. È importante, dunque, fronteggiare le difficoltà di sindaci e amministratori locali e chiaramente di tutti gli altri soggetti attuatori. Penso soprattutto alle situazioni dei piccoli Comuni, che devono anticipare le spese per realizzare le opere. Sono 70.000 i Comuni sotto i 5.000 abitanti coinvolti in altrettanti progetti finanziati appunto dal Piano. Così come penso alle difficoltà delle imprese chiamate a lavorare nei cantieri, che devono fare i conti, ad esempio, con i rincari dei materiali. Questo Governo -come dicevo prima - sta lavorando proprio su questo: snellire le procedure e semplificare i processi eliminare alla radice tutti gli ostacoli, che impedivano già prima e impediscono ancora oggi la messa a terra delle risorse dei nostri territori. Su questo punto c'è oggi l'impegno di tutto il Governo e di tutta la maggioranza. vorremmo che dall'opposizione non si levasse una voce di critiche solo strumentali e propagandistiche. Non è possibile che vi sia qualcuno che tifa contro gli interessi dell'Italia. Ripeto il PNRR è una partita che non può avere colori politici. Noi riteniamo che debba esserci una necessaria flessibilità. E su questo punto sosteniamo convintamente l'operato del Governo, che sta concretamente lavorando per modificare i progetti, che erano stati studiati e presentati - come dicevo prima - quando il quadro era completamente diverso rispetto a quello attuale. Riteniamo si debba fare di tutto per utilizzare al massimo i fondi messi a disposizione, quelli a debito e non, per favorire la modernizzazione e la crescita del Paese. Sosterremo, senza sé e senza ma, il Governo e il lavoro puntuale e approfondito che sta facendo il signor Ministro per l'utilizzo dei fondi del PNRR. Non possiamo e non dobbiamo sprecare alcun euro. Questa partita la giochiamo - come dicevo prima - per l'Italia e per gli italiani. Al PNRR però va fatto un tagliando, con tutto il rigore e l'attenzione necessari - come prima ha spiegato bene - in maniera costruttiva e responsabile. A differenza di chi agita la bandiera della propaganda, preferiamo lavorare a testa bassa e, con il Governo, grazie al lavoro del Ministro in Europa, preferiamo intraprendere la strada della revisione seria del PNRR, che è un'operazione che avrebbe fatto chiunque al nostro posto. L'azione del Governo italiano si sta dimostrando efficace, perché è stata scelta l'opzione cosiddetta giuridica. In altre parole, ogni richiesta è avanzata non come pretesa, ma come istanza legittima. È un approccio - secondo noi e secondo me - intelligente, pragmatico e sicuramente vincente, signor Ministro. Il PNRR è uno strumento che deve unire e non può dividere. La rimodulazione del PNRR è una partita che non può essere strumentalizzata politicamente, perché i protagonisti sono i territori e, quindi, tutti i nostri cittadini. In gioco non ci sono solo il Parlamento o il Governo, ma ci sono i Comuni, le Province, le Regioni e quindi tutti i cittadini e tutte le imprese. Se seduti ai banchi del Governo ci foste voi, oggi sareste voi ad evidenziare la necessità della rimodulazione del Piano. Quindi, basta sprecare fiato contro gli interessi dell'Italia! Crescita, occupazione, PNRR: il Governo Meloni sta lavorando bene, per dare risposte concrete agli italiani. Tra l'altro, qualche giorno fa la CNN ha giudicato positivamente l'operato del Governo.

giudica positivamente l'informativa del ministro Fitto e sostiene il suo operato e quello dell'intero Governo.

difficoltà e girano voci su una difficoltà nell'attuazione di questo Piano straordinario, che per il nostro Paese è fondamentale, come ho già avuto modo di dire. Le prime responsabili sono

Un altro elemento è quello della transizione ecologica. Avete posto una questione sul 2035 e sul 2050. Faccio però un esempio banale.

ha detto bene la Commissione europea: gli stadi li facciano le società di calcio, perché non si possono pagare miliardi i giocatori e poi chiedere soldi pubblici per realizzare gli stadi. Intervengano loro da questo punto di vista, e su questo sono perfettamente d'accordo.

caso, almeno leggendo le cose che sono state scritte anche dal Presidente dell'ANCI, i Comuni mi sembrano molto disponibili alla discussione e al confronto per accelerare l'attuazione del PNRR. In sostanza - e chiudo - ciò che

in apertura del mio intervento - è importantissimo per lo sviluppo e per ridurre le disuguaglianze del Paese. Se, alla fine del processo, avremo invece aumentato le disuguaglianze, in questo caso sarà stato un grande fallimento.

sul PNRR italiano si giocano due partite vitali, per cui bisogna dosare con grande attenzione le parole e rifuggire, ove possibile, dalle tentazioni polemiche o strumentali. La prima partita riguarda il futuro dell'Italia. È una *chance* storica, un treno che non passerà mai più sulla possibilità di sciogliere ritardi e nodi strutturali del sistema Paese, e questo con l'aggravante che altri quel treno lo stanno prendendo, scavando un solco incolmabile in termini di competitività. La seconda riguarda il destino dell'Europa. Sul Next generation EU si gioca l'idea di un'Europa come progetto di mutuo soccorso tra gli Stati membri e l'impegno per far avanzare il processo di integrazione. Per queste ragioni, signor Ministro, apprezziamo la sua rinnovata disponibilità a venire a riferire in Parlamento; così come apprezziamo la chiarezza con la quale ha espresso il suo punto di vista e con la quale, soprattutto, ha confermato la centralità del Parlamento e il suo pieno coinvolgimento nelle scelte degli obiettivi da rimodulare e sul monitoraggio del procedimento. Certamente è vero: tra missioni, componenti, priorità trasversali, investimenti e riforme propedeutiche l'Europa ha dato agli Stati membri un piano di regole di non semplice attuazione; così com'è vero che non sarebbe corretto gettare sull'attuale Governo l'intera croce delle difficoltà e dei problemi che lei prima ha enunciato. Con la stessa franchezza, però, signor Ministro, bisogna dire che le scelte compiute dal Governo e dai partiti che lo sostengono non hanno aiutato a migliorare la situazione. situazione. Oggi appare chiaro che chiudere in modo così brusco la passata legislatura avrebbe comportato talune criticità, perché, per quanto possa essere ordinato il passaggio di consegne, sempre di passaggio di consegne si tratta. Allo *spoils system* all'interno delle strutture ministeriali, con la riforma della *governance* di cui ci ha parlato proprio nel suo intervento, avete anche aggiunto quello delle strutture di missione. Mesi e settimane senza garantire continuità, con gli interrogativi legati alla rinegoziazione del Piano, diventano ovviamente un problema se si è chiamati a fare un percorso che richiede ferrea disciplina sui tempi e sulle scadenze. Allo stesso modo, la riforma della *governance* che - come lei stesso ha detto - si è completata oggi, non offre risposte adeguate sulle criticità emerse nei primi mesi di attuazione, e non basta introdurre premi di produttività per i dirigenti comunali. Serve semmai introdurre un sistema sanzionatorio per tutti quegli organismi che non rilasciano le autorizzazioni e ostacolano o frammentano il procedimento amministrativo. Questo sarebbe di grande aiuto soprattutto al Sud, dove, troppo spesso, il diverso colore politico tra un Comune e un ente superiore fa sì che certi progetti vengano bloccati o rallentati per strategia politica. Quello che più ci preoccupa, tuttavia, è come vi state relazionando con l'Europa in questa fase, innanzi tutto sui tempi. L'Europa chiedeva agli Stati membri di presentare eventuali richieste entro il 30 aprile: noi non solo non facciamo questo, ma dalla maggioranza arrivano anche posizioni diverse tra chi parla di semplice rimodulazione dei progetti e chi invece invita a rinunciare a parte delle risorse; tra lei, signor Ministro, che parla di spostare alcuni progetti sul Fondo di sviluppo e coesione, e i Presidenti delle Regioni - con in testa Fedriga - che dicono che quelle risorse non si toccano. Prendiamo atto, signor Ministro, con sincero apprezzamento, delle sue parole di oggi sulla rimodulazione degli interventi, in particolare per gli asili nido, con l'impegno a mantenere le risorse per il Mezzogiorno. E vogliamo pensare che questa sia la posizione di tutto il Governo Non può sfuggire che la rottura del vincolo del 40 per cento delle risorse a favore delle Regioni meridionali sarebbe un atto politico gravissimo, innanzi tutto perché, se l'Italia è la principale beneficiaria delle risorse europee, è proprio per via dei ritardi strutturali delle Regioni meridionali; in seconda battuta perché si cristallizzerebbe a questo punto e per sempre il divario sociale ed economico fra le due parti del Paese. Per noi tutto quello che è stato dato deve essere speso. Bisogna attrezzare il Paese nella sfida complicata e affascinante di un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale. Bisogna rimuovere i tanti ostacoli che hanno impedito al Sud di esprimere le sue potenzialità per la per la crescita complessiva del Paese. Bisogna ricucire il quadro sociale perché, senza asili nido, parlare di denatalità e del miglioramento del ruolo delle donne diventa soltanto vuota e insopportabile retorica. È dunque arrivato il momento delle responsabilità, il momento di essere pronti per governare il Paese, e su questo impegno, signor Ministro, ci troverete pronti a offrire la nostra capacità e competenza per il raggiungimento del traguardo che - come lei ha ben detto - è quello del giugno 2026.

che sembra volto a tenere il PNRR lontano dal logorio del dibattito politico quotidiano. È un tentativo apprezzabile, che noi abbiamo provato a condividere, pur dai banchi dell'opposizione, quando si è trattato di affrontare e di confrontarci sul decreto della *governance*. Le diamo atto con piacere e con convinzione del fatto che essere qui a riferire in Parlamento sul PNRR è un modo per condividere i contenuti di quel Piano, esattamente come lei in quell'occasione ci diede atto di aver tenuto come opposizione un atteggiamento differente, attraverso un voto di astensione e delle proposte. di Carlo Calenda su Industria 4.0; penso alla richiesta di un'unica unità di missione per quanto riguarda Italiasicura. Questo è stato il modo di Azione-Italia Viva-RenewEurope col quale confrontarci sulla *governance* e dare il nostro contributo.

chi ha gridato al fatto che il PNRR andrebbe interamente riscritto; chi ha provato a scaricare su Comuni, Province e Regioni la responsabilità del non fatto; chi addirittura si è alzato per dire che i soldi sono troppi, dopo anni di razionalizzazione e di difficoltà nel reperire le risorse. Noi invece cogliamo questa occasione per ribadire la nostra posizione, che non è mai cambiata: per noi il PNRR va attuato, le risorse vanno spese integralmente e le riforme vanno approvate subito, perché non sono meno importanti degli investimenti. Non c'è una terza via, non c'è tempo da perdere, anche perché avete avuto dal Parlamento il via libera sul decreto *governance;* siete in carica da sei mesi; dovrete contrattare con la Commissione europea le modifiche a cui lei faceva cenno; avete il compito di stendere il Repower EU e quindi è una vostra responsabilità raggiungere gli obiettivi del semestre. Per questo dico che non ci sono alibi e il tempo delle verifiche sta per terminare. La *deadline* è quella del 30 giugno, data entro la quale dovrete dimostrare di aver conseguito gli obiettivi previsti e spero che voi siate in grado di farlo esattamente come il Governo che vi ha preceduto. che vi ha preceduto. Se occorrerà poi adeguarsi alle modifiche della Commissione, credo che questo vada fatto, Ministro. Forse Forse di polemiche con la Commissione europea ce ne sono state anche troppe: ora è il tempo di mettere a terra questi investimenti e di mantenere con l'Europa e con la Commissione europea un rapporto di dialogo. Per questo ben venga la decisione di non opporre resistenza allo stralcio dello stadio di Venezia e dello stadio di Firenze, che sono progettualità degli enti locali che possono trovare soluzioni differenti. È meglio utilizzare quelle risorse per le riqualificazioni urbanistiche delle città, come sottolineato prima da Matteo Renzi. *(Applausi)*. Troppo spesso si è discusso di PNRR in modo molto generico; lei ha provato ad entrare nel merito di alcuni nodi e io vorrei tornare su quei punti. Il primo è quello degli asili nido. Su questo penso che sia molto importante portare a termine la missione 4 del Piano, perché dentro quella missione ci sono scelte fondamentali per le nuove generazioni: non solo gli asili nido, ma penso che i decreti attuativi della riforma degli istituti tecnici superiori (ITS) o dell'istruzione professionalizzante siano alcuni punti fondamentali della messa a terra del PNRR. scelta, poi, che avete avanzato di spostare alcune progettualità dal PNRR alle politiche di coesione ve ne dovete assumere la responsabilità e rispetto a essa noi individuiamo alcuni rischi, perché proprio lei qualche giorno fa illustrava - e lo ha richiamato anche quest'oggi - il fatto che solo il 34 per cento della spesa della coesione (126 miliardi) è andato a buon fine. buon fine. Se questo sia un modo per accelerare, quindi, lo scopriremo strada facendo, perché ad oggi le politiche di coesione non hanno dato risultati brillanti. Accanto al tema degli asili nido c'è anche un'altra questione che mi sta molto a cuore e che lei, Ministro, ha toccato solo in parte: quella delle infrastrutture. Ci ha confermato difficoltà per alcune opere,

sullo Stretto. Ciò nonostante, il nostro atteggiamento è assolutamente costruttivo e responsabile. Noi sempre, anche dai banchi dell'opposizione, tifiamo Italia. Siamo consapevoli che la crescita di questo Paese dipenderà dalla vostra capacità di mettere a terra gli investimenti del PNRR e che la stima e la credibilità del Paese dipenderanno in buona parte dal successo dell'operazione. Le facciamo quindi moltissimi auguri e ancora una volta confidiamo che lei possa, quando a maggio dovrà rappresentare lo stato di avanzamento del PNRR, darci delle buone notizie, perché ne abbiamo veramente bisogno.

Devo constatare che il dibattito intorno al PNRR si sta facendo molto più intenso in questi ultimi sei mesi che non nel periodo precedente, forse perché il Piano è stato concepito in un momento storico particolare della vita italiana, in una stagione di Governi multiformi di salvaguardia, che ha fatto sentire tutti compartecipi, ma allo stesso tempo esenti da reali responsabilità. Proprio la prima versione del Piano, per certi versi improvvisata, è la genesi di tutte le questioni delle quali oggi discutiamo. Probabilmente la discussione in passato è stata annacquata proprio per l'assenza di una reale contrapposizione, col paradosso che un serrato confronto come quello di oggi è utile alle forze politiche, al Governo, ma soprattutto ai cittadini, che traggono informazioni, conoscenze e occasioni di valutazione. È un Piano che comprende investimenti di entità mai vista in passato come lei sottolineava - per certi versi troppo ambizioso rispetto agli obiettivi temporali prefissati; finanziamenti assegnati all'Italia non per merito di qualcuno come una falsa narrazione ci voleva far credere - ma grazie a criteri oggettivi: il maggior calo del PIL nel periodo della pandemia, la crescita della disoccupazione, il numero degli abitanti in rapporto alla popolazione europea; finanziamenti, quindi, che devono essere distribuiti su tutto il territorio nazionale, Ministro, perché sono stati destinati proprio per superare le condizioni più svantaggiate in cui versano alcune Regioni del Sud. Sarebbe paradossale se qualcuno pensasse com'è stato anche proposto - di impiegare queste risorse più cospicuamente al Nord, aumentando il *gap* infrastrutturale e lasciando pure i cittadini del Sud indebitati per il futuro. È un Piano che mette a disposizione grandi risorse, ma il prezzo di questa grandezza è la responsabilità. Ecco di cosa parliamo, Ministro: non è una scelta la sua, ma è una responsabilità. Lo fa in una posizione davvero critica e delicata - lo capisco e partiamo dalla posizione critica, e non tanto per i tre obiettivi di cui ha parlato, non centrati e che sta cercando di risolvere, sbloccando la terza rata.

Il nostro Paese storicamente ha difficoltà a spendere, nei tempi stabiliti, le risorse assegnate per gli investimenti: lo so bene da sindaco di una città e anche, per un periodo, da Presidente della Commissione sui fondi di coesione di ANCI. La situazione attuale dei fondi di coesione

e questa percentuale si è ottenuta solo grazie ad opere già avviate con la legge obiettivo. In 34 mesi abbiamo speso circa 10 miliardi di euro e nei prossimi mesi che ci separano, cioè nei restanti 44 mesi, dovremmo spendere circa 220 miliardi di euro. Il dato allarmante è che si è praticamente spenta in Italia - quasi del tutto negli ultimi dieci anni - la capacità di spesa da parte della pubblica amministrazione, forse proprio a causa dell'abitudine, anche negli ultimi periodi, di erogare risorse in conto esercizio per l'aumento dei salari bassi e per il reddito di cittadinanza, e non effettuare investimenti in conto capitale. Poi c'è l'altro problema, che è quello dell'*iter* delle opere pubbliche. Paesi dell'Unione europea l'Italia è la penultima, prima della Grecia. Per realizzare un'opera pubblica di 100 milioni di euro si arriva fino a quindici anni. Lei ha parlato adesso di mettere in salvo dei progetti che da qui a tre anni dovranno essere completamente realizzati, per una spesa complessiva enorme. Tutto ciò è stato aggravato da norme introdotte anche di recente: basti pensare al regolamento che, insieme al codice degli appalti del 2016, ha contribuito a dilatare i tempi di oltre il 50 per cento, a causa delle varie procedure per il controllo delle offerte inserite nello stesso, cosa risolta nel nuovo codice approvato dal Governo Meloni che introduce, al contrario, un principio della fiducia. fiducia. L'ultimo tema riguarda la carenza del personale. Per moltissimi anni gli enti locali hanno dovuto scontare il blocco del *turnover*, che ha impedito le assunzioni, favorendo così non solo l'invecchiamento del personale in servizio, ma anche una desertificazione degli uffici,

scade nel 2026 e non è un caso che il suddetto decreto assunzioni contempli anche la possibilità di stabilizzare il personale precario, che è già formato. È una posizione delicata, la sua, signor Ministro, anzi direi scomoda politicamente, perché richiede coraggio per correggere e recuperare una situazione difficilissima.

L'obiettivo è spendere tutte le risorse messe a disposizione; di spenderle bene, però, per progetti utili e necessari, visto che una parte di questi finanziamenti - come sappiamo - andrà restituita e graverà sui nostri figli e nipoti. Oggi c'è l'esigenza di far ripartire il Paese e di sostenere il PIL nei prossimi anni; c'è anche un obbligo etico, però, ed è quello di rispondere alle sfide che ci attendono come appartenenti alla comunità globale, riguardo ad esempio ai cambiamenti climatici. Uno sviluppo sostenibile non solo deve promuovere la conservazione delle risorse per le generazioni future, ma deve anche sollecitare attività produttive compatibili con gli usi futuri. Signor Ministro, lei è venuto qui in Parlamento e non si è sottratto al confronto, chiedendo la collaborazione di tutti. Lo ha fatto con signorilità, con un comportamento istituzionale, evitando polemiche rispetto al passato. Ha chiarito che, per incassare dall'Unione europea, non sono sufficienti solo le riforme e gli atti formali, ma occorre la anche dimostrazione di concreta e misurabile capacità di spesa. Ha proposto soluzioni di buon senso sullo stato di attuazione e i risultati sono - quelli che dicevamo - dei fondi di coesione. È più che mai necessario mettere mano alla *governance* centralizzando la capacità di intervento. Lei ha recepito le richieste dei Comuni, delle Province e delle Regioni, che hanno approvato questa rimodulazione della *governance* nella Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali. E ha spiegato che non sarebbe possibile in altro modo creare quelle giuste interazioni funzionali e, al tempo stesso, inserire alcune opere del PNRR nei programmi supportati dai Fondi sviluppo e di coesione. Sarà infatti necessario togliere dal PNRR alcune opere - lo ha detto prima - che non hanno alcuna possibilità di rispettare la scadenza del 2026, per inserirle nella nuova programmazione dei fondi strutturali e dei fondi di coesione, che hanno scadenze più lunghe. Le somme recuperate da questo travaso andranno ad alimentare, rendendolo uno strumento più credibile, il nostro programma Repower, che la Commissione europea ha intrapreso come ulteriore tassello, con l'obiettivo di porre fine alla dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili della Russia e affrontare la crisi climatica. Signor Ministro, lei ha fatto benissimo a coinvolgere in tutto questo le nostre aziende pubbliche, come diceva prima - hanno una forte capacità organizzativa e gestionale come ENI, Enel, Ferrovie, Snam, Terna, perché sicuramente ci consentiranno di recuperare buona parte del tempo perduto realizzando le grandi infrastrutture necessarie. ha fatto tutto questo e lo ha fatto molto bene, ma la responsabilità non si ferma solo all'aspetto gestionale: essa riguarda il coinvolgimento sui temi etici che sono alla base del Piano, a cui noi aderiamo e per cui ci indebitiamo. Sono sei missioni, quelle del PNRR, che ci riconducono però a tre fondamentali princìpi: la transizione ecologica e la mobilità sostenibile; la salute e il benessere delle persone; l'istruzione e l'inclusione sociale. Sono tre princìpi rivolti agli uomini e alla loro vita, soprattutto a quella delle generazioni future in un'ottica di sostenibilità. L'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono semplicemente delle azioni al servizio di questi primi concetti così importanti. Impiegheremo circa 85 miliardi per la transizione ecologica e non possiamo mantenere un comportamento tiepido e distaccato su questo tema, quasi fosse una moda o una tendenza del momento, come sostiene Non possiamo sperare che cambino gli equilibri in Europa solo per rivedere queste politiche, perché, a prescindere dalle maggioranze, non sarà possibile ormai svincolarsi da questi obiettivi. Il clima sulla terra è sempre stato soggetto a mutamenti climatici, oggi, per la prima volta nella storia del pianeta, stanno aumentando a velocità pazzesca, senza precedenti. La spiegazione è semplice e dipende dalle innovazioni tecnologiche prodotte negli ultimi Per migliaia di anni abbiamo avuto solo tre innovazioni tecnologiche per il *confort* termico: nelle case, per esempio, prima il camino, poi il vetro alle finestre e infine la stufa. Il XIX secolo è stato la culla delle tecnologie, che si sono affermate nel XX secolo, fino all'uso esagerato e non rispettoso dei giorni nostri, che produce ovviamente un inquinamento con velocità esponenziale. Cinquanta miliardi sono le tonnellate di gas serra che vengono emesse ogni anno nell'atmosfera,

Un aumento così rapido provocherebbe l'aumento di eventi atmosferici estremi. Su questi argomenti l'Italia non può essere il fanalino di coda in Europa. Non serve dire che possiamo incidere poco sulle emissioni globali, perché abbiamo una responsabilità etica. Noi siamo l'ottava potenza economica, ma soprattutto abbiamo un primato culturale nel mondo e dobbiamo stare in prima fila riguardo a questi temi. Incentivare queste politiche vuol dire creare un vantaggio competitivo per le nostre imprese, che saranno più innovative nel futuro, anziché restare per ultime su posizioni di retroguardia. Sono molte le cose che si potrebbero fare, anche attraverso lo strumento dell'affidamento in concessione con gare internazionali. Lei lo sa: si possono rigenerare molti siti abbandonati, circa 90.000 chilometri quadrati chilometri quadrati di aree industriali dismesse, che rappresentano il 3 per cento del territorio nazionale. Si può agire con opere di rigenerazione urbana, bonificare i tanti siti inquinati, mettere in sicurezza il territorio, fare un complesso progetto di approvvigionamento idrico, con ottimizzazione delle risorse e creazione degli invasi nell'intero territorio nazionale. Ha tanto lavoro da fare, signor

Questo è l'approccio che le abbiamo indicato proprio qui in Aula, quando abbiamo parlato del decreto-legge PNRR. Occorre visione e occorre rimodulare il PNRR con una concezione complessiva, insieme alle parti sociali e alle parti politiche di tutto il Paese.

il mese di maggio. Ci aspettavamo qualche informazione in più, visto che leggendo gli articoli di stampa ci si lancia in determinate dichiarazioni, soprattutto da parte della maggioranza (come abbiamo notato). Alcuni interventi vengono tolti, perché mettevano a rischio la terza rata; però oggi lei non ci ha riferito come verranno sostituiti (ancora non si sa). sa). E di chi è la responsabilità politica? Lei ha citato un decreto interministeriale; ci sarebbe piaciuto sapere anche di chi è la responsabilità politica e chi è che ha individuato i progetti da inserire nel PNRR (decreto (decreto interministeriale del 22 marzo 2022). Ci sarebbe piaciuto saperlo, tutto qua; ma non è stato detto e non ci è dato saperlo oggi. Io però credo che questa ricognizione stia creando qualche preoccupazione e qualche cortocircuito, nella maggioranza e nel Paese.

è una carenza di monitoraggio sia del PNRR che della politica di coesione. Mancano 18.000 progetti al monitoraggio: vuol dire che non si ha idea del reale avanzamento del Piano. Stessa considerazione per il piano complementare al PNRR e per la politica di coesione generale. Il collettore dovrebbe essere la banca dati unitaria, che però non parte, non funziona, i dati non arrivano.

se la piattaforma centrale non funziona, come facciamo ad avere il quadro complessivo dei progetti che vengono attuati, che possono essere attuati oppure no? Su questo, quindi, io non aspetterei maggio, ma comincerei ad intervenire, visto che alcune proposte sono già arrivate, anche da ANCI, proprio sul decreto PNRR. Sono Sono arrivate tantissime segnalazioni: difficoltà di accesso, continue modifiche alle pagine, i Comuni non riescono ad inserire i dati, i manuali operativi necessari tardano ad arrivare. Parliamo ora, invece, dell'altra preoccupazione che ha sollevato oggi questa informativa, quella sulla quarta rata e su alcuni progetti che potrebbero essere non completati. Oggi noi ci saremmo aspettati delle rassicurazioni da parte sua, soprattutto sul raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati per sbloccare la quarta rata, in particolare per i progetti che riguardano la costruzione di nuovi asili nido. nido. Questa misura era già stata prorogata. La scadenza era prevista per dicembre e poi è stata spostata al 31 marzo, data che era stata prevista prima. A poco più di un mese dal termine, però, nonostante le proroghe, i problemi non sono stati risolti. Per il nostro Paese rappresenterebbe veramente una perdita notevole quella di uno dei progetti di infrastrutture sociali più importanti per contrastare il grave problema della denatalità, un problema che voi avete sollevato proprio in questi giorni. Parlare di voler affrontare la denatalità senza un occhio di riguardo ed un'attenzione maggiore per la realizzazione di tutti i progetti inseriti, non solo di quelli retrospettivi, me lo sarei aspettato da questo Governo. Noi, però, non possiamo permetterci, come italiani e come Paese, di rinunciare a investimenti determinanti per la crescita, l'emancipazione sociale e la lotta alle disuguaglianze. Anche in virtù dei progetti che possono essere a rischio all'interno del PNRR, voglio fare una riflessione e rivolgere una raccomandazione, soprattutto per alcune tipologie di progetti che per me hanno una importanza, anche perché vengo dalla Sicilia. Stiamo parlando dei progetti dedicati all'ammodernamento della flotta per il traghettamento sullo stretto di Messina che, nel giro di pochi anni, avrebbe consentito e consentirebbe spostamenti più rapidi e sicuri, con mezzi a minore impatto ambientale. Queste misure sono previste all'interno del PNRR. a tutela della continuità territoriale non viene oggi messa in discussione, per fortuna, neanche dalla incapacità dei vari uffici, ma è gravemente pregiudicata, a nostro avviso, dalla propaganda per la costruzione di un ponte da 15 miliardi, che non si sa se e quando sarà mai realizzato. *(Applausi)*. Noi non vogliamo neanche immaginare che il Governo ipotizzi di tagliare risorse certe per necessità impellenti allo scopo di perorare promesse irrealizzabili, giocando sulla pelle dei cittadini siciliani e calabresi. Questa è la raccomandazione che facciamo: salvare tutti i progetti utili per l'Italia, al di là delle difficoltà, con quell'approccio che lei ha già espresso durante la sua informativa, e di cui la ringraziamo. Si tratta di un approccio che vede coinvolte tutte le forze politiche le forze politiche e le forze sociali del Paese. Abbiamo già visto che sono iniziati i primi lavori della cabina di regia, il 19 e il 20 aprile, anche se nei comunicati stampa alcune forze sociali si sono lamentate e l'hanno visto più come un tavolo interlocutorio che un confronto. Ci auguriamo che i prossimi tavoli siano invece più dedicati al confronto e utili per il territorio. Come MoVimento 5 Stelle siamo sempre disponibili al confronto. Avevamo proposto un tavolo, che a quanto pare è stato rifiutato, ma saremo sempre disponibili qui, in Assemblea, in Commissione e ovunque il Governo ritenga opportuno e necessario affrontare i problemi

Soprattutto diamo un consiglio alle minoranze: è meglio forse spostare un po' il tiro, perché su questo argomento vedo poca sostanza, rispetto all'ottimo lavoro che il Governo sta facendo.

dal Governo giallorosso, con il presidente Conte. In questi casi, infatti, quando si vuole alimentare la crescita, prima bisogna individuare quali sono le opere quali sono le opere che di fatto possono creare investimenti e sviluppo per il Paese e, in base alle opere, chiedere le risorse a disposizione. Invece qui è stato chiesto il massimo delle risorse e poi, nella classica mentalità italiana piatto ricco: mi ci ficco! - si è inserito dentro tutto il possibile e l'immaginabile, non curandosi di quello che effettivamente poteva essere utile o meno al Paese *(Applausi)* e soprattutto di quali potevano essere i risultati e la messa a terra, a livello realistico, del Piano.

L'intervento andava in quella direzione e sarebbe assurdo, con tutte le difficoltà che ci sono, andare ad indebolire la *governance*. Bisognava certamente dare una mano per rafforzarla e infatti il Governo ha puntato a migliorare l'organizzazione della struttura della pubblica amministrazione, con la stabilizzazione del personale e con il consolidamento delle strutture. È stata riorientata - almeno questo è l'intendimento del Governo - l'offerta privata su alcuni bandi che magari sono andati deserti. Si vogliono mettere in campo delle garanzie statali proprio a sostegno delle aziende, molte delle quali magari sono anche un po' in difficoltà per questioni legate al mercato di oggi. A proposito di mercato, sì, è vero che i mercati internazionali ci dicono che gli investimenti sono cruciali per la tenuta dei nostri conti pubblici, ma è proprio per questo motivo che è necessario di fatto un intervento del Governo per rendere realistico il piano; è proprio funzionale a quella che è un'esigenza a livello nazionale e anche di mercato.

per noi va bene perché poi il risultato finale è stato che tutta la maggioranza ha detto e ribadito più volte che è giusto puntare, come anche lei, Ministro, ha detto oggi, sui progetti per i quali i finanziamenti possono essere spesi entro il 2026, che è la razionalità del Piano. Non è dire qualcosa fuori dalla dalla norma, ma semplicemente affermare una cosa ovvia. Se però siete contenti così, va bene, anche perché la crescita di lungo termine di lungo termine non dipende dalla quantità della spesa, ma dalla qualità degli investimenti

deve sobbarcarsi nel corso del tempo. Questo è un atteggiamento molto pragmatico e razionale - perdonatemi anche un minimo di orgoglio personale - di chi comunque, al Nord, del pragmatismo ha fatto una virtù, con risultati che si sono anche visti nel tempo.

cui noi dobbiamo sempre guardare come faro nelle nostre politiche, hanno chiesto solo ed esclusivamente il fondo perduto e non i prestiti. Anche questo è un dato che ricordiamo: noi,

che riceve un finanziamento che però poi non rispetta le scadenze volute dal Piano, l'Italia deve rimborsare il finanziamento e poi terminare le opere a proprie spese. È quindi evidente e chiaro che il Governo vuole rimodulare, essere certo degli interventi, puntare sulle risorse che verranno spese. È un modo di governare di buon senso che adotterebbe chiunque. Io mi chiedo, alla luce di queste richieste, di questi interventi e chiarimenti, come sia possibile fare polemica. Sì, lo è per chi non ha argomenti.

le questioni che riguardano la *tranche* di dicembre e soprattutto 3 dei 55 obiettivi. Volevamo però rassicurare il Ministro che su quei temi, grazie alle nostre interlocuzioni, ma anche al dibattito sui giornali, sapevamo che si sarebbe arrivati per quanto riguarda gli stadi, le concessioni portuali e il tema del teleriscaldamento. Quello che noi invece vorremmo sapere, signor Ministro - e glielo vogliamo chiedere con grande nettezza e con grande chiarezza sui prossimi obiettivi, ma soprattutto quali sono i progetti che lei intende spostare sul Fondo di coesione. Ha parlato con le Regioni? Quali sono le criticità? Quali sono i progetti sul REPower (2,7 miliardi), su cui già altri Paesi stanno presentando i loro progetti? Sulle case della salute andiamo avanti o ci fermiamo? Sul tema degli asili nido, che sono un obiettivo fondamentale per la conciliazione di famiglia e lavoro, andiamo avanti o ci fermiamo? Lei ha detto che su questo - e ha buttato la palla in tribuna - ci informerà in una successiva occasione: ma noi l'informativa l'abbiamo chiesta proprio per questo. Allora, visto che lei non ci ha risposto, proviamo a mettere in fila e ad articolare le nostre preoccupazioni, indicando anche qualche proposta, così la prossima volta magari ci risponde su questi temi molto ben precisi. Parto dalla prima questione. Quali sono i progetti che intende spostare sui fondi di coesione? Lo chiedo perché, come sa meglio di me, non è proprio facile nell'interlocuzione con le Regioni, in Conferenza Stato-Regioni, trovare progetti, chiaramente garantendosi più flessibilità soprattutto sui tempi, anche perché le Regioni hanno già fatto la loro programmazione, hanno individuato gli obiettivi con le comunità locali, con le associazioni di categoria. Proprio quell'interlocuzione di cui lei parlava prima

al contrasto alla povertà energetica e al sostegno alle comunità energetiche, prima veniva ricordato il fatto che mancano alcuni decreti attuativi per la spinta sulle energie rinnovabili. rinnovabili. Signor Ministro, un pezzo di lavoro lei lo ha già fatto, perché sta incontrando le aziende partecipate di Stato; con Eni ed Enel sta discutendo di quali progetti presentare sul REPower. Qual è la difficoltà a venire qui in Parlamento e a condividerli con noi nelle Aule in cui si dà l'indirizzo politico? Perché non ci racconta di quei progetti? Vogliamo sapere, ad esempio, se a Catania, dove c'è già una fabbrica enorme per la produzione dei pannelli fotovoltaici, siamo in grado di costruire una filiera produttiva italiana, facendo un pezzo di politica industriale sui pannelli fotovoltaici. Se ne può fare un'altra? È uno dei progetti che rientra nel REPower EU? Vorremmo discutere tra di noi, scelga se in Commissione o qui in Aula, ma abbiamo il diritto e il dovere di poterlo fare anche qui. Siccome ci sono delle interlocuzioni in Aula, vorremmo capire anche noi quali sono i progetti sul REPower EU: immagino che lo vorrebbe sapere anche la Commissione europea, visto che accumuliamo ritardi su ritardi. Non c'è solo il tema della *governance*, ma anche della possibilità di andare avanti da questo punto di vista. Le nostre preoccupazioni si addensano anche sui temi che riguardano la salute. Abbiamo fatto una battaglia per garantire più di 20 miliardi nel PNRR, per metterne 7 per le case della salute. Io vengo da una Regione, la Lombardia, che ha patito più di altre il Covid nella fase iniziale e abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che cosa ha voluto dire una scarsità di presenza di Rete sui servizi territoriali, un modello molto ospedalocentrico, con difficoltà a garantire quelle cure a bassa intensità che sarebbero state necessarie in quella fase per intervenire tempestivamente e non arrivare a portare pazienti già compromessi nelle terapie intensive dei nostri ospedali. Vogliamo tornare indietro al 2019 e fare finta che non sia successo niente? Le case della comunità possono essere l'*hardware*

Gettiamo la spugna davanti a uno degli interventi principali all'interno del PNRR, atteso da tempo dalla nostra comunità, sui temi su cui siamo più sensibili come quello della sanità? La situazione è analoga per quanto riguarda gli asili nido: è ancora più grave, perché il messaggio sarebbe sbagliato, ovvero gettare la spugna su uno dei servizi essenziali nella prima fase della formazione, dell'educazione della prima infanzia. Lo dico perché è uno di quegli interventi che incrocia anche obiettivi trasversali che affrontiamo, quali il tema dei divari di genere e quello dell'occupazione femminile: il 30 per cento rimane un obiettivo ancora lontano, motivo per cui le chiediamo e le richiediamo di presentare quelle linee guida proprio per andare

Come si fa a presentare, da una parte, un programma da 7 miliardi per contrastare la denatalità e, dall'altra, pensare di smantellare gli asili nido che sono una delle prime infrastrutture che permettono di conciliare lavoro e professione e di coniugare le aspirazioni delle nostre famiglie e delle donne in particolare?

previsti 900 milioni già dal passato Governo da poter utilizzare per la spesa corrente per l'assunzione proprio di maestri e maestre per gli asili nido, tra l'altro anche in deroga ai limiti assunzionali; quindi, non ci sono proprio scuse da questo punto di vista. Aggiungo un altro tema che ha a che fare con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Noi facciamo giustamente il nostro lavoro di opposizione, denunciamo puntualmente le cose che non funzionano, ma abbiamo l'interesse che funzionino, perché è una grande occasione. Siamo andati in Europa, abbiamo lavorato per costruire le condizioni perché si intervenisse sul debito comune, perché si affermassero gli Eurobond, che era qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa: sono stati stanziati 190 miliardi.

con ANCI e nell'interlocuzione con la Commissione, a ragionare sul fatto che, raggiunto un certo limite percentuale di asili nido già aggiudicati, si possa avere magari qualche giorno in più anche oltre la data del 30 giugno, perché i Comuni stanno lavorando bene. i Comuni hanno già assegnato 31 dei 40 miliardi, e addirittura hanno impegnato quasi 18 miliardi delle risorse loro assegnate, proviamo a fare come ha fatto il precedente Governo proprio su iniziativa del Partito Democratico, che in quei progetti di rigenerazione urbana sopra i 15.000 abitanti ha stanziato risorse *ad hoc* per andare a coprire anche quei progetti che erano inseriti nella lista degli idonei, ma non finanziati. Ecco, proviamo anche con la Commissione a contrattare spazi di flessibilità per aiutare quei Comuni che hanno presentato progetti sulla rigenerazione urbana, sull'edilizia scolastica, sui parchi: progetti interessanti, già ritenuti idonei, che però non hanno finanziamento. Insomma, prima di alzare bandiera bianca su una grande occasione di sviluppo e crescita del nostro Paese, vediamo di fare di tutto perché quei soldi vengano spesi bene e vengono dati a quelle amministrazioni comunali che hanno dimostrato di saperli spendere bene, nell'interesse delle nostre comunità.

innanzitutto ringraziare il ministro Fitto perché la sua presenza costante e continua in quest'Aula e anche durante i lavori

Il PNRR è stato approvato nel 2021, quando le priorità dell'Italia e dell'Europa erano un po' diverse rispetto a quelle che ci sono oggi. allora uscendo dal Covid e il PNRR è nato proprio per rilanciare la nostra Nazione, l'economia e la coesione nelle nostre Regioni. Chi ha scritto questo piano si è concentrato maggiormente sul portare a casa quattrini dall'Europa che sul ragionare e focalizzare quali erano i progetti da finanziare ed è questo forse il *vulnus* di questo Piano. Se c'è una parte di Piano che è a fondo perduto

generare PIL, da dare valore aggiunto al sistema Italia, proprio per giustificare l'impegno di spesa ulteriore che l'Italia dovrà affrontare per coprire la quota capitale e la quota interessi. Concentrandoci troppo sui quattrini da portare a casa, come dicevo prima, dovevamo anche pensare che

quella soluzione, a nostro modo di vedere, doveva essere ponderata nel miglior modo possibile e doveva essere applicata a progetti che dessero valore e creassero PIL per la nostra Nazione.

In questo contesto e per consentire una forte accelerazione nella realizzazione degli interventi in esso previsti, il Governo infatti ha messo in campo il decreto-legge n. 13, che è uno strumento che è stato pensato e studiato proprio per attenuare i grandi impedimenti che ostacolavano la concreta realizzazione dei fondi del PNRR. Analizzato e approvato in quest'Aula e poi alla Camera dei deputati, ha visto il coinvolgimento di tutte le forze politiche nel corso del suo *iter* parlamentare. in legge, contribuirà a far sì che le amministrazioni attuatrici portino a compimento il loro obiettivi entro le scadenze prefissate. Le parole d'ordine, fondamentali per arrivare a compimento, sono state snellimento, semplificazione, flessibilità e politica osmotica delle risorse, proprio per quei progetti che rischiano di non essere portati a termine. Questa legge ha introdotto delle novità molto importanti su tutta una razionalizzazione della *governance*, volta a fornire una maggiore efficienza. La nuova struttura di missione PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assumerà il coordinamento strategico per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano e degli obiettivi e i traguardi concordati a livello europeo. Vengono rafforzati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di inerzia e di ritardo, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze da parte delle amministrazioni attuatrici, che al contempo potranno, a loro volta, riorganizzare le unità di missione dedicate all'attuazione del Piano. Presidente, chiedo al senatore Alfieri quante volte nei due anni precedenti ha portato in discussione i temi che poc'anzi ha portato in quest'Aula, perché queste sono

Infine, questo provvedimento ha affrontato i temi della transizione e della sovranità energetica, che possiamo definire l'argomento più importante e attuale per l'Italia. La programmazione aggiornata e soprattutto il capitolo relativo al Repower EU si sviluppano lungo due assi: il primo riguarda il coinvolgimento delle grandi partecipate dell'energia (Eni, Enel, Snam e Terna). Forse uno Stato stratega, che avesse - come dicevo prima - studiato prima i progetti e poi chiesto le risorse, avrebbe coinvolto in modo più presente e puntuale queste importanti società che rappresentano lo Stato italiano. Sono stati introdotti chiarimenti e semplificazioni per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare gli impianti che consentiranno la produzione di energia *green,* per il rilascio delle autorizzazioni e per l'installazione di impianti di impianti fotovoltaici, impianti eolici e di accumulo energetico e impianti agrofotovoltaici. Gli sforzi ora si dovranno concentrare nell'ottenimento dalla Commissione europea di ulteriori forme di flessibilità per indirizzare al meglio i fondi del PNRR, i fondi strutturali e i fondi di coesione su progetti che abbiano ricadute significative per il nostro sistema produttivo e sociale e per dotare il nostro Paese di una solida politica industriale che permetta alle imprese italiane di cogliere le opportunità date dalla duplice transizione ecologica e digitale. Come più volte ribadito dal Governo e dalla maggioranza, il nostro obiettivo è che nemmeno un euro dei fondi PNRR vada perduto, ma anzi si traduca in maniera efficace in un beneficio per la nostra Nazione. Questa non è la sfida del Governo Meloni, di questa maggioranza parlamentare, di un singolo partito o di una coalizione; è la sfida dell'Italia. Lo ribadisco rivolgendomi soprattutto a chi in questi ultimi mesi, in tema di PNRR, sta alimentando una narrazione tendenziosa e negativa per l'Italia, imputando a questo Governo colpe e ritardi che non trovano alcun riscontro nella realtà dei fatti. La stessa Commissione europea ha riconosciuto l'esigenza di modificare il percorso originariamente tracciato. Il Governo Meloni da mesi sta lavorando a stretto contatto con la Commissione, proprio nell'ottica di risolvere i principali problemi strutturali di questo Piano. Per tutti noi, come recentemente ribadito anche dalla presidente Meloni, il PNRR è un'opportunità che il Governo non si lascerà sfuggire. Proprio per queste ragioni, alle facili e inutili polemiche a cui abbiamo assistito in questi primi sei mesi di legislatura, rispondiamo con il nostro impegno continuando a lavorare nell'ottica di rimodulare il PNRR fino a giugno 2026. L'Italia e gli italiani vogliono portare a compimento questi progetti perché rivestono un'importanza strategica per la ripartenza della nostra Nazione. Il ministro Fitto ha ricevuto un incarico non facile, ma che sta portando avanti con grande responsabilità, ed è proprio questa grande responsabilità che ci dovrebbe unire e non dividere. La responsabilità è quella di scrivere, grazie a queste risorse per l'Italia, il futuro delle prossime generazioni. La mia non è retorica ma - ahimè - una dura realtà, perché se sbaglieremo qualcosa o non sfrutteremo al meglio questa grande opportunità, il danno sarà per tutti. il ministro Fitto. Fratelli d'Italia sarà sicuramente al suo fianco per realizzare al meglio il PNRR, per l'Italia e per gli italiani.

di Potenza-sezione civile». Con ricorso depositato il 23 maggio 2022, il tribunale ordinario di Potenza-sezione civile ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 febbraio 2022, ha dichiarato l'insindacabilità - ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - delle dichiarazioni rese da Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento civile

Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 23 marzo 2023. Nella seduta del 5 aprile 2023, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione. Chiedo al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Franceschini, se intende intervenire.

Signor Presidente, colleghi e colleghe, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge: non si tratta di un mero principio presente tra i diritti fondamentali della Costituzione, trascritto in ogni aula di giustizia, per poi non essere applicato. Esso rappresenta proprio il cardine dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo sempre adottato una linea chiara e coerente relativamente all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il quale non deve essere inteso come privilegio della politica, ovvero come scudo attraverso il quale ripararsi da qualsivoglia azione giudiziaria. Tutti i cittadini, infatti, senza alcuna distinzione, nel momento in cui vengono chiamati a processo, hanno il dovere di parteciparvi al fine di esercitare correttamente il loro diritto di difesa. Coerentemente con il suddetto assunto, anche in questo procedimento abbiamo votato in senso opposto rispetto alle formulazioni della Giunta, poiché, a nostro modo di vedere, il legame temporale e il legame fattuale fra le dichiarazioni *intramoenia* ed *extramoenia* non sembravano necessariamente attestati, e in tal modo la prerogativa *ex* articolo 68 della Costituzione non avrebbe non avrebbe operato pienamente, come previsto sulla base degli elementi individuati dalla Corte costituzionale in relazione all'applicabilità dell'articolo. Ora, però, ci troviamo in una fase successiva, ovvero quella relativa al sindacato sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. ho detto in premessa, abbiamo votato in maniera contraria rispetto alle deliberazioni della Giunta, ma l'Assemblea, che è sovrana, ha deciso di ribadire le conclusioni emerse dall'esame in sede decentrata. caso il discorso non attiene più a logiche politiche, perché la questione è la difesa dell'istituzione che rappresenta i cittadini. Quando l'Assemblea del Senato prende una decisione, salvi casi imprevisti ed eccezionali, quella decisione Sarebbe illogico privare il Senato della possibilità di costituirsi in giudizio a difesa delle proprie prerogative, per mezzo di un voto espresso proprio da quei soggetti che *in primis* dovrebbero tutelarlo. Per tali ragioni esprimo il voto favorevole da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere in un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Potenza-sezione civile. *(Segue la votazione).*

Signor Presidente, mi permetta di fare un brevissimo accenno al fatto che io ho frequentato le scuole superiori a Giarre e quindi mi sento partecipe della visita oggi dei miei corregionali, che mi ricordano tanto gli anni della gioventù. *(Applausi)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sento il dovere oggi di intervenire per segnalare una vicenda triste, ma anche piena di speranza. È la storia del tragico incidente È la storia del tragico incidente accorso a Leonardo Lotto, ventiquattro anni, di Aosta, che, a causa di un tuffo sbagliato su una spiaggia di Melbourne in Australia, per una tragica trama del destino, è ora paralizzato dal collo in giù. Leonardo però è un giovane coraggioso e forte. «Muoverò le braccia, camminerò ancora» ha detto, usando una frase a noi già conosciuta: *whatever it takes*, a qualunque costo. Voglio richiamare questa vicenda per continuare ad esprimere la mia vicinanza a questo giovane coraggioso e alla sua famiglia e per dare il giusto merito a chi è stato capace, in un Paese straniero, con lingua, cultura e procedure diverse dalle nostre, di sostenere la famiglia di Leonardo in quei primi tragici, devastanti giorni, che nessun genitore vorrebbe mai vivere. Mi riferisco alla nostra rete consolare e diplomatica e, in prima linea, alla console generale di Melbourne, Anna Pappalardo, che, malgrado le difficoltà derivanti dalla mancanza di personale, ha fatto squadra ed operato con determinazione, competenza e velocità, affinché i genitori e lo stesso Leonardo ricevessero assistenza mentre era in ospedale e per il pericoloso e complesso viaggio di rientro in Italia. Sono le istituzioni che si attivano e agiscono nell'interesse supremo dei cittadini italiani all'estero. Allo stesso tempo, però, non posso non segnalare al ministro Tajani che purtroppo, sia in Australia che in Nuova Zelanda, i nostri consolati hanno bisogno di attenzione da parte del Ministero, per assicurare il personale di ruolo e a contratto locale necessario per svolgere i loro servizi. Occorre adeguare livelli salariali ed altre condizioni di impiego. Signor Presidente, mi permetta di fare un ultimo accenno a Leonardo Lotto, che era in Australia per completare l'ultimo semestre del suo corso di laurea, iniziato alla Bocconi e proseguito presso l'Università di Singapore. Purtroppo il destino ha voluto che i flutti dell'oceano nascondessero un banco di sabbia, dove si è tragicamente concluso il suo tuffo. Un giovane che, con tanta speranza ed impegno, si accingeva a completare un eccellente corso di studi, per poter portare il suo contributo nel mondo del lavoro. Un bellissimo esempio delle eccellenze del nostro Paese. Malgrado le sue condizioni Leonardo, in un *post* sui *social network* sorride e, usando la famosa frase di Mario Draghi, dice: «Non posso che guardare avanti. Mi aspetta un nuovo viaggio, che sarà doloroso e molto duro. A volte cadrò, ma alla fine mi rialzerò e continuerò a combattere, facendo tutto ciò che serve. *Whatever it takes*». Signor Presidente, è questa la speranza che possiamo trarre da questa triste vicenda. *Whatever it takes*: non quello di Mario Draghi, ma quello di Leonardo Lotto. Nei momenti difficili dobbiamo rialzarci, con determinazione e forza. Lo dobbiamo a Leonardo, ai milioni di italiani all'estero e a quelli che ci chiedono assistenza per i diritti anche al di là dei nostri confini.

dopo una triste agonia. Tutti i colleghi, gli amici e coloro che la conoscevano si sono stretti intorno al mondo della psichiatria, una realtà che è stata, di fatto, lasciata a se stessa dopo la chiusura degli dopo che tutta una massa di persone, che evidentemente hanno dei problemi di grave natura psichiatrica, si sono riversate sulla psichiatria territoriale. purtroppo, non ha strumenti, se non il TSO, per gestire questo grande numero di persone, che gira in maniera libera per le nostre strade, che può andare addirittura a cercare un dottore, in questo caso una psichiatra, fino al punto di aspettarla sotto la sede di lavoro per poi aggredirla. La psichiatria ha bisogno di norme e di strutture che diano la possibilità di esercitare su questi soggetti pericolosi un controllo. Per farlo, occorre uscire da quella ideologia che, ahimè, ha ritenuto sufficiente chiudere gli OPG per risolvere un problema. Mentre effettivamente la libertà personale va salvaguardata, perché è un bene assoluto, occorre anche individuare nuovi strumenti normativi e sanitari per gestire soggetti non in grado di intendere e di volere. Soprattutto, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, non è più tollerabile procrastinare un intervento normativo in materia.

Signor Presidente, è con grande commozione che vorrei ricordare in quest'Aula una nostra collega, in questo Senato che è scomparsa nei giorni scorsi a Rosario in Argentina, dove viveva. Mi riferisco alla senatrice Mirella Giai, che è stata qui cinque anni in rappresentanza del Maie e che è stata sicuramente una protagonista importante degli italiani in Argentina. È morta all'età di novantatré anni. Era figlia del comandante Giai, emigrato in Argentina e rientrato nel 1943 per combattere la guerra partigiana nelle Brigate Garibaldi del Piemonte. Successivamente, di nuovo emigrò con la famiglia a Rosario. Lei fu impegnata profondamente nell'associazionismo. Assieme a Filippo Di Benedetto operò nel periodo della dittatura di Videla, in collaborazione con il console dell'Italia Enrico Calamai, nell'assistenza all'espatrio di centinaia di italiani, che furono sottratti così al destino dei *desaparecidos*. Alle elezioni del 2006 si candidò al Senato e fu eletta: la realizzazione del suo sogno, come la realizzazione del sogno di tanti italiani che all'emigrazione e all'italianità nel mondo hanno dedicato la loro esistenza. la loro esistenza. L'ho conosciuta, anche se in quegli anni ero alla Camera dei deputati. Abbiamo avuto un'intensa collaborazione nell'ambito dell'interparlamentare e sono veramente stato conquistato dal carisma di questa donna, dalla sua serietà, dal suo impegno e dalla sua concezione di una politica fatta al servizio della comunità nazionale. Credo che questo fosse in fondo lo spirito con cui, durante gli anni della mia Presidenza della Camera dei deputati, istituimmo la figura dei rappresentanti degli italiani all'estero: fu soprattutto l'onorevole Tremaglia che fece quella battaglia, come Ministro per gli italiani nel mondo. Quell'esperienza, come tutte le esperienze, ha luci e ombre, ma sicuramente, se ha tante luci, esse si devono alle figure più eminenti e più significative. Vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare il presidente La Russa, che si è associato nei giorni scorsi con una bellissima dichiarazione alla comunità italiana di Argentina per questa scomparsa. Mi inchino alla memoria di Mirella e credo sia molto significativo che agli italiani di Argentina arrivi la solidarietà direttamente dall'Assemblea del Senato della Repubblica. Ringrazio il presidente Casini per aver svolto questo intervento e per aver doverosamente ricordato la senatrice Giai. Senatore Casini, anche io in quella legislatura la ricordo. La Presidenza tutta si associa quindi al sentimento di cordoglio per i familiari e per tutta la comunità